Il relatore, senatore Guerrieri Paleotti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi Signor Presidente, signori Ministri, senatrici e senatori, vorrei ricordare innanzitutto che con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza il Governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza, presentato ad aprile, unitamente agli obiettivi programmatici, questi ultimi anche in considerazione delle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea. L'operazione di aggiornamento del DEF serve pertanto a tracciare i confini della manovra e delle misure che conterrà la legge di bilancio, che va approvata entro il 20 ottobre. Insieme alla Nota di aggiornamento al DEF 2017, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo, già autorizzato con le risoluzioni di approvazione del DEF 2017. In estrema sintesi, si può affermare che i dati contenuti nella Nota di aggiornamento delineano due andamenti entrambi positivi: l'economia italiana consolida la sua espansione e cresce più del previsto; dall'altro, il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, che ha un particolare valore strategico per tutta una serie di ragioni che chiarirò in in seguito, diminuisce già da quest'anno ed è previsto continui a diminuire nel corso dell'intero periodo coperto dalla Nota di aggiornamento. Veniamo innanzitutto al quadro macroeconomico, che si presenta particolarmente favorevole: l'economia mondiale si è rafforzata in tutte le aree del mondo, compresa l'area dell'euro, che è cresciuta con particolare intensità grazie alle politiche monetarie fortemente espansive della Banca centrale europea. L'economia italiana ha sfruttato in positivo questo andamento ciclico favorevole e si prevede crescerà dell'1,5 per cento nel 2017, avendo già acquisito 1'1,2 per cento nella prima metà di quest'anno. Siamo al decimo trimestre consecutivo in cui il PIL dell'Italia mostra il segno positivo e la ripresa in corso rappresenta la fase di espansione più lunga degli ultimi due decenni. Rispetto alle passate fasi di ripresa, tuttavia, la sua dinamica è ancora lenta e continua a risultare inferiore alla media dei nostri *partner* europei, anche se la distanza si sta riducendo. Resta comunque il dato molto positivo quest'anno dell'accelerazione della crescita, accompagnata da una relativa diffusione della dinamica di espansione, dall'industria manifatturiera ai servizi privati. Una crescita più elevata e stabile è, certo, il frutto del quadro internazionale e europeo più favorevole e della grande creazione di liquidità generata dalle politiche monetarie non convenzionali messe in atto da tutte le banche centrali dell'area più avanzata ultima, in ordine di tempo, la BCE - dal marzo 2015. Ma tra questi fattori determinanti - va subito aggiunto - figurano a pieno titolo le riforme e le politiche messe in campo in Italia negli ultimi anni le misure portate avanti dal Governo in questo ultimo anno, quali il rilancio degli investimenti e le misure per ristabilire il regolare funzionamento del sistema bancario. Secondo il quadro tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento, l'economia italiana crescerebbe dell'1,2 per cento nel 2018 Le proiezioni del quadro programmatico indicano un proseguimento più favorevole, invece, della dinamica di espansione nel 2018 e 2019 a tassi pari a quanto raggiunto quest'anno, ovvero l'1,5 per cento Le previsioni di consenso a livello europeo e internazionale sono più caute e individuano nei due anni successivi al 2107 un rallentamento della crescita di 0,2-0,3 punti percentuali sia per l'area euro sia per la nostra economia. Come è noto, non è facile esprimere un giudizio su queste proiezioni programmatiche, visti l'elevata incertezza e i rischi geopolitici che incombono sul prossimo futuro. Si può dire, però, che per il 2018 il quadro economico internazionale si manterrà favorevole e, quindi, potrà continuare a sostenere la dinamica di espansione dell'economia italiana secondo quanto previsto nella Nota di aggiornamento. Per il 2019, invece, il previsto rallentamento a livello europeo e internazionale fa sì che solo una decisa ripresa della domanda interna italiana potrà consentire di raggiungere l'obiettivo di crescita del quadro programmatico. In questo caso, l'elemento trainante potrebbe essere rappresentato dagli investimenti, sia pubblici sia privati. Nelle previsioni del Governo dovrebbero accelerare sia le spese in macchinari e attrezzature, che beneficerebbero degli incentivi del piano Industria 4.0, sia quelli residenziali, gli acquisti di case, che dovrebbero crescere con un relativo maggiore dinamismo. A questo riguardo va fatto notare che, di recente, vi sono indicazioni di un rafforzamento strutturale della domanda interna di macchinari e provengono per quest'anno, secondo l'ISTAT, dagli indicatori derivanti dalle indagini sulle imprese e dalle rilevazioni dirette sui giudizi e le aspettative degli imprenditori. Per quanto riguarda la manovra di bilancio, essa sarà - com'è noto - di circa 20 miliardi di euro complessivi, gran parte dei quali serviranno per eliminare gli aumenti dell'IVA previsti nel 2018, che costano circa 15,6 miliardi. Circa 10 miliardi verranno dal maggior *deficit* messo in programma nel 2018 e altrettanti da nuove misure per circa 0,5 punti di PIL (ripartiti in 0,2 punti sul fronte dei tagli di spesa e 0,3 con nuove entrate), soprattutto con una nuova stretta all'evasione, dalla fatturazione elettronica tra i privati ad altre misure allo studio. Per le spese si tratterebbe, in sostanza, di nuovi interventi sui Ministeri e l'amministrazione centrale. È evidente che le risorse così reperite restano limitate e dovranno essere pertanto concentrate su pochi mirati obiettivi, che vengono indicati nella Nota di aggiornamento rispettivamente in alcuni interventi per il rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati, altri interventi sull'occupazione, a partire dall'annunciato intervento sul costo del lavoro con sgravi contributivi per sostenere l'occupazione giovanile, e nelle politiche per l'inclusione sociale, attraverso il rafforzamento di misure di contrasto alla povertà. A questo riguardo, vorrei sottolineare che porre al centro dell'azione di politica economica i giovani e la loro occupazione è di per sé un gesto molto significativo per un Paese che - come sappiamo - forma dei giovani ad elevata competenza e poi li esporta senza riuscire a importarne di altrettanto pregiati. Vengo al quadro di finanza pubblica. Complessivamente la Nota di aggiornamento presenta un quadro tendenziale migliore di quello atteso nel DEF di aprile, anche grazie a un quadro macroeconomico - come ho prima ricordato - più favorevole. In particolare, la Nota stima che l'indebitamento programmatico netto nel 2018 sarà pari all'1,6 per cento rispetto al 2,1 per cento nel 2017, grazie alla ripresa ciclica e alla riduzione della spesa per interessi. Allo stesso tempo, il Governo programma di accrescere l'indebitamento netto nel 2018 di oltre 0,5 punti rispetto al suo andamento tendenziale. Va sottolineato che limitare l'aumento del disavanzo pubblico all'1,6 per cento del PIL, pur essendo probabile che la Commissione europea avrebbe accettato fino all'1,8 credo rappresenti il segno concreto che il Governo intende accelerare la riduzione del *deficit* di bilancio negli anni seguenti, come prospettato nella Nota di aggiornamento. L'indebitamento netto passerebbe in effetti all'1,2 per cento nel 2019 e allo 0,2 per cento nel 2020, raggiungendo a questo punto il sostanziale pareggio di bilancio. Anche per il saldo strutturale il miglioramento programmato per il prossimo anno è inferiore a quello indicato nel DEF di aprile. Il *deficit* strutturale sarà ridotto nel 2018 dello 0,3 per cento rispetto allo 0,8 per cento Un dato particolarmente significativo è - secondo il programma della Nota - che il rapporto tra *stock* di debito e PIL diminuirebbe già da quest'anno,

Alla fine dell'orizzonte di programmazione, il rapporto si attesterebbe al 123,9 per cento. Va ricordato, a questo proposito, che per il 2015 l'ISTAT, nella revisione operata dei conti, ha giù registrato una leggera riduzione del debito, che è passato al 131,5 per cento del PIL (dal 131,8 per cento dell'anno precedente). Questi risultati di riduzione dello *stock* di debito sul PIL sarebbero ottenuti grazie sia ad avanzi primari crescenti nel tempo, sia ai proventi delle privatizzazioni,

Al riguardo, va sottolineata la sorpresa negativa di questi mesi, che è venuta proprio dall'inflazione, mantenutasi molto al di sotto dei valori attesi, in seguito sia alla tendenza alla rivalutazione dell'euro, che ha ridotto il costo dei beni importati, sia alla dinamica estremamente modesta di aumento delle retribuzioni. Si potrebbe obiettare che la riduzione del rapporto tra *stock* di debito e PIL valga inizialmente solo pochi decimali. Ma va ribadito che la discesa del rapporto, per quanto lieve, è altamente significativa, perché tale inversione di tendenza, dopo anni di crescita ininterrotta, è il segnale atteso sia dai mercati, sia da Bruxelles. L'altro motivo per cui è importante che nel 2017 il rapporto fra debito e reddito nazionale sia più basso che nel 2016 che nel 2016 e continui a diminuire è che a fine ottobre la Banca centrale europea farà sapere come intende ridurre gli acquisti di titoli di Stato, dopo averne comprati per circa 2.000 miliardi di euro, di cui quasi 300 miliardi emessi da Roma. La fine del *quantitative easing* (QE) è un dato certo, mentre i suoi tempi e le sue modalità sono ancora da definire. Anche per questo la nostra economia, tenuto conto che tra qualche mese comincerà la stagione elettorale, dovrà mettersi nelle condizioni di presentarsi pienamente credibile all'appuntamento della fine del QE. Va altresì considerato che mantenere un tale percorso credibile, pur se graduale, di consolidamento del debito avrebbe effetti positivi anche sul ruolo potenziale che potremmo giocare, come Paese importante dell'Unione europea, nel negoziato che si sta per aprire, dopo le elezioni tedesche, per un ripensamento e un auspicabile rilancio del processo di integrazione. Per riassumere, gli obiettivi di finanza pubblica della Nota di aggiornamento del DEF sono coerenti con la volontà del Governo di bilanciare sostenibilità fiscale e sostegno alla ripresa economica e appaiono compatibili con l'impostazione prefigurata dalle istituzioni europee, volta a utilizzare più ampi margini di discrezionalità nel valutare il rispetto delle regole europee, anche al fine di assicurare la cosiddetta *fiscal stance*, ovvero un risultato di politica fiscale complessiva per l'area dell'euro che sia appropriata al contesto di crescita in corso. Il Governo, nel confermare l'impegno a ridurre il disavanzo e lo *stock* di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL nel 2017 e negli anni seguenti, ha presentato alle Camere anche la relazione al Parlamento, redatta ai sensi ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale ha chiesto alle stesse Camere l'autorizzazione a deviare dal percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine (il pareggio di bilancio in termini strutturali), in modo da conseguire il pareggio di bilancio nel 2020, slittando di un anno rispetto a quanto previsto ad aprile nel DEF. Com'è noto, l'ordinamento nazionale prevede che eventuali scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali e previa autorizzazione approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, indicando, nel contempo, il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine. Tale piano può essere altresì aggiornato qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo decida di apportarvi delle modifiche. A fronte di tale ultima necessità, si è giustamente ritenuto opportuno richiedere alla Commissione europea, pur rimanendo entro i parametri e i vincoli comunitari, un rinvio temporale e un rallentamento del percorso di consolidamento dei conti pubblici e, quindi, di usufruire di risorse aggiuntive e di tutti i margini a disposizione per predisporre una manovra di bilancio che preveda misure per la crescita e il sostegno dei redditi dei cittadini. Su tale linea, tra l'altro, si sta muovendo la stessa Commissione europea - come ho già messo in rilievo - in ragione della necessità di dare maggiore respiro e slancio alla crescita dell'area dell'euro e dell'Unione europea nel suo insieme. Il quadro presentato nella Nota di aggiornamento e nella relazione è dunque quello definito in questi mesi anche con la Commissione europea, anche se il giudizio europeo arriverà - come sappiamo - solo con la bozza di *budget* che andrà inviata entro il 15 ottobre. Per concludere, credo sia importante sottolineare il doppio obiettivo che il Governo consegna alla prossima legge di bilancio: una finalità più ambiziosa sul versante della crescita e un deciso avvio della riduzione del rapporto debito/PIL. I dati contenuti nella Nota di aggiornamento - come ho cercato di argomentare in questa mia relazione - offrono una conferma che la direzione intrapresa sia quella giusta. Tutto ciò è positivo, ma non vuol dire che ci si possa accontentare. Va fatto di più e l'imperativo è quello di ulteriormente accelerare la crescita e renderne visibili gli effetti in termini di nuova consistente occupazione, soprattutto dei giovani. Ma crescere di più e più rapidamente vuol dire rilanciare a medio termine produttività e progresso tecnico della nostra economia. È una strada lunga - come sappiamo - che non ha scorciatoie e non è certo una scorciatoia imboccare il percorso di una aumentata spesa pubblica in disavanzo. Lo abbiamo già fatto in passato, con risultati sempre negativi e deludenti. L'accelerazione della crescita è un'operazione da accompagnare con un'accorta politica di bilancio, che prepari il terreno a nuove e incisive riforme, anche perché il prossimo anno - come ho già detto - col graduale esaurirsi del *quantitative easing*, i conti pubblici devono essere posti in assoluta zona di sicurezza. Solo in questo modo non saremo più visti, con una percezione che naturalmente va giudicata eccessiva, come un Paese a rischio in Europa. È dunque un momento importante quello che caratterizzerà l'ultima manovra di bilancio della legislatura, quella che precede le elezioni della prossima primavera. Il rischio da evitare è disperdere il dividendo della maggiore crescita, facendo nuovamente lievitare il debito. La percezione di aver superato la fase di crisi deve in realtà spingerci a portare avanti ulteriori politiche che riducano il debito e irrobustiscano la crescita. l'unica via per superare e metterci alle spalle vecchi modelli e metodi che ci hanno sempre penalizzato in passato. Ricordo che l'Annesso alla Nota di aggiornamento reca la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo. Ai sensi del richiamato articolo 6, commi 3 e 5, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del Documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta;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

non è così scontato che i Governi siano così prudenti nel fare previsioni ottimistiche. Altre buone notizie sono l'accelerazione dei flussi turistici e dell'esportazione di beni, la graduale ripresa degli investimenti - di certo ancora bassa, ma è sicuramente una ripresa l'impennata della produzione e delle aspettative nel comparto dei beni strumentali. Continua la crescita dell'occupazione: oltre 23 milioni di unità.

per l'assunzione a tempo determinato. I dati più recenti indicano un ulteriore rafforzamento della crescita nella seconda metà dell'anno. Vi sono una rinnovata fiducia degli operatori e un sensibile miglioramento nel settore del credito. Il debito pubblico ha finalmente invertito la tendenza e si prevede per il 2018 la discesa al di sotto del 130 130 per cento. Si è lavorato per una finanza pubblica sostenibile e favorevole alla crescita, in un clima di riforme strutturali per la competitività e la fiducia, e costruendo con l'Europa una nuova *governance* per affrontare nuove sfide. Le audizioni che abbiamo svolto questa settimana ci hanno confortato. L'Ufficio parlamentare di bilancio, sulla base di una valutazione complessiva delle previsioni del Governo, ha deciso di validare lo scenario programmatico,

La Corte dei conti, che ha espresso parere favorevole sulla recente revisione dei dati di contabilità nazionale, dà conto di un biennio 2015-2016 su molti fronti migliore rispetto alla precedente rendicontazione. Inoltre, un cospicuo afflusso di dati congiunturali documenta come si sia di fronte a una ripresa superiore alle previsioni. Il miglioramento dei conti pubblici, conseguito dall'Italia negli ultimi anni, consente, già nel 2018, una forte riduzione dell'indebitamento netto tendenziale e un rafforzamento dell'avanzo primario. Nel 2020, azzerato il disavanzo, l'avanzo primario raggiungerà il 3,5 per cento del prodotto. La Corte dei conti sottolinea anche alcuni aspetti problematici, ma conclude con una valutazione positiva. lo stesso vale per la Banca d'Italia. giustamente non si è soffermato. Voglio soffermarmi sul capitolo V della Nota di aggiornamento che riguarda le riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. europea. È un capitolo molto importante che illustra le riforme adottate e il loro stato di attuazione dopo la pubblicazione del Programma nazionale di riforma ad aprile 2017, aprile 2017, nonché le raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea e come ad esse si stia rispondendo attraverso l'azione di Governo. Alla luce degli obiettivi posti dall'Unione europea, che per la prima volta pongono l'accento su una intonazione di bilancio a supporto della crescita, si raccomanda all'Italia una politica fiscale basata sulla revisione della tassazione sulla prima casa, sulla riforma del catasto e sul rafforzamento della fatturazione e dei pagamenti elettronici. Negli altri ambiti, la Commissione richiama alla necessità di procedere nel cammino di riforma per la modernizzazione del Paese.

porre un accento, perché è un aspetto che è stato sempre sottolineato negli ultimi anni: gli enti locali sono un nuovo volano per gli investimenti e per una ripresa locale e veloce. L'altro L'altro aspetto riguarda il catasto, ove si dice che nell'ambito del processo di revisione del sistema catastale di classificazione degli immobili sono state implementate alcune attività finalizzate alla costruzione di un'anagrafe immobiliare integrata, gestita interamente una nuova piattaforma, che integra le informazioni relative al territorio con quelle relative ai proprietari. Questo è veramente importante, perché consentirà un approccio molto diverso per tutta la finanza locale.

dalle relazioni programmatiche sulle spese d'investimento per ciascuna misura di spesa. Non ho tempo a disposizione per entrare nel merito di questi due ampi fascicoli, ma vorrei sottolineare alcune curiosità,

perché riguarda la realizzazione dei lavori di completamento del banchinaggio, drenaggio e raccordo stradale della diga di Molfetta. Questo è solo per dire che ci sono informazioni dettagliate, estremamente utili per noi che proveniamo dai territori; informazioni

Vi limitate ad elencare una serie di presunti successi guardando a dati che certamente risentono del clima di ripresa generale che investe l'Europa, ma che non possono e non devono alimentare facili illusioni rispetto allo stato reale della nostra economia. Sappiamo bene che i segnali positivi sono in larga parte ascrivibili all'azione della Banca centrale europea, come ci ha più volte ricordato anche la Banca d'Italia, e non alle scelte di questo Esecutivo; scelte sempre più politiche e che di certo non incoraggiano i segnali di ripresa. Politica è, ad esempio, la scelta, che considero drammatica, di definanziare in modo progressivo la spesa pubblica per la salute. La Nota di aggiornamento, infatti, non introduce alcun correttivo alle previsioni di finanziamento per la sanità,

le conseguenze sono pesanti: aumento della spesa privata e crescente rinuncia alle cure. Occorre prendere atto subito che le politiche degli ultimi anni hanno fallito e cambiare rapidamente direzione, facendo diventare la vertenza per la salvaguardia del *Servizio sanitario nazionale* (SSN) perché si arrivi ad investire nella salute, si riducano le diseguaglianze, partendo dall'abolizione del superticket di 10 euro sulla ricetta, siano sostenuti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) e si rafforzi il personale sanitario, con particolare attenzione alle zone marginali, a quelle montane e a quelle o con maggiore difficoltà di mobilita interna. Politiche sono altresì le scelte di impoverimento degli enti locali. All'interno della Nota di aggiornamento vengono elencate le risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio delle loro funzioni. Anche in questo caso, spiace dirlo, quanto fatto non è abbastanza. Province e Città metropolitane versano in condizioni drammatiche, con le prime che risentono significativamente degli effetti negativi prodotti da una legge incompleta (la legge Delrio), che non tiene nemmeno conto di principi all'interno dei quali vengono riconosciute aree con specificità, in particolare le Province interamente montane.

molti dei quali in dissesto economico, ed evitare che a pagare il prezzo più grande della crisi siano i soggetti più deboli. In ultima analisi, servono misure di buonsenso, soprattutto in una situazione in cui la crisi finanziaria è frutto di scelte sbagliate che hanno deliberatamente impoverito questi enti.

questo documento risulta comunque, come i precedenti, del tutto inattendibile. Predisporre documenti inattendibili determina, a fine anno, l'aumento del debito pubblico. Signor Ministro, non è possibile che alcuni esponenti del Governo dichiarino sui giornali che il Governo ha tagliato il debito pubblico. Questo Governo è il primo produttore mondiale di debito pubblico. Nel mese di luglio ha sfondato quota 2.300 miliardi con un aumento, rispetto al mese precedente, di 18,6 miliardi, 82 miliardi in più rispetto al primo gennaio 2017. Siamo ad un aumento di debito pubblico di 304 milioni al giorno.

Naturalmente, il debito pubblico determina l'aumento delle tasse. Il DEF stabilisce che dal 2017 al 2020 avremo un aumento delle tasse di 81 miliardi. sommando l'incremento delle tasse che è ben certificato: si passa dai 786 miliardi del 2016 agli 867 miliardi del 2020. non ci sono riduzioni di spesa perché oltre a pagare gli interessi sul debito pubblico, c'è la spesa pubblica che cresce. Infatti, il DEF prevede che nel 2020 avremo 30 miliardi di spesa pubblica in più. Naturalmente, il Paese, oltre al problema del debito pubblico, ha il problema della disoccupazione. I livelli di disoccupazione in Italia sono tra i più elevati d'Europa e la riduzione della disoccupazione, come

giovani ogni anno, soprattutto giovani laureati, lascino il nostro Paese per cercare di fare fortuna nel resto del mondo. Sono giovani laureati la cui formazione è costata al cittadino italiano oltre 165.000 euro. Il DEF cosa che un capitolo della prossima legge di bilancio riguarderà misure per la competitività e l'innovazione. In questo ambito sono compresi interventi sul costo del lavoro volto ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Per questo capitolo spendiamo la bellezza di 338 milioni di euro nel 2018, cioè spendiamo la produzione del debito di un giorno. Facciamo 300 milioni di debito in un giorno e spendiamo per incentivare l'occupazione giovanile 338 milioni

Bisognerebbe fare innovazione e ricerca. Ebbene, le risorse riservate agli investimenti nel DEF, nell'anno 2018, ammontano a 300 milioni. Infine, chiudo parlando del Fondo sanitario nazionale. Voi siete furbi che più furbi non si può. Ogni anno, sui documenti, stanziate qualche miliardo in più.

queste somme sul bilancio, ma non le impegnate e non le erogate. I tagli cumulati sul Servizio sanitario nazionale negli ultimi tre anni ammontano a 10,5 miliardi.

e che spendo sul tema della sanità, non solo per l'ovvio dovere d'ufficio che mi compete, ma anche per raccogliere e far camminare, nel sentiero stretto di cui ci ha parlato il ministro Padoan, preoccupazioni, attese e proposte che da questo mondo ci pervengono. È vero, il Paese va meglio, ma non va abbassata la guardia. Prudenza e responsabilità: il sentiero è comunque stretto e c'è spazio per poche e qualificate scelte. Questo è il messaggio della NADEF: una crescita che va sostenuta e che richiede attenzione e prudenza.

anche trasformando le difficoltà che questo comporta in grandi opportunità per il Paese. A cosa mi riferisco? I numeri di questi anni parlano da soli: la spesa sanitaria cresce sì in valore assoluto, ma si riduce la sua incidenza sul PIL. La spesa sanitaria pubblica *pro capite* in Italia è mediamente inferiore di un terzo rispetto a quella dei Paesi I disavanzi regionali per anno sono scesi dai 6 miliardi del 2006 a poco più di un miliardo, così quantificato nel 2016. \*\*\*Dietro questi freddi numeri c'è però un mondo molto complesso, un mondo che, come dicevo, ha trasformato delle difficoltà in opportunità. Guardate al nuovo modello di *governance* dei livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale (Stato-Regioni); in questi anni sono cresciuti procedure e modelli di controllo e programmazione della spesa, di verifica della spesa, di verifica e di erogazione dei LEA, di informatizzazione. ha certamente contribuito a restituire elementi di efficienza ed efficacia al sistema. Ma, dietro a questi numeri, ci sono anche altri fattori,

*turnover*, nell'emergere e nell'affermarsi di aree sempre più vaste di precariato all'interno del Servizio Così come ci sono - diciamolo, perché è responsabile dirlo - aree grigie di equità e di universalismo nell'erogazione dei vecchi e dei nuovi LEA; questo lo dicono un po' tutti gli istituti di ricerca che lavorano in materia.

che stanno dentro il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La stima al momento è ancora ambigua perché mancano atti, ma è ragionevole pensare che si tratti di 500-600 milioni Così come si riproporranno anche quest'anno le modalità di contributo delle Regioni a statuto ordinario all'equilibrio della finanza pubblica.

che probabilmente per la quota ancora da pagare, che non è indifferente, andrà in transazione. C'è però un problema; le Regioni hanno già iscritto nei bilanci, così come prevedeva la legge, l'intero importo delle cifre. cifre. Solo la somma di tutto questo, in un mero ragionamento contabile, ci fa capire come l'incremento della spesa non si riesca a coprire. a coprire. Se è vero che dobbiamo recuperare efficienza ed efficacia del sistema, dobbiamo fare attenzione

che il nostro impegno, proprio in quel sentiero stretto, ma comunque responsabile e rigoroso, affinché vengano riviste alcune previsioni di spesa sanitaria, nasca da una semplice convinzione: una buona sanità

Ricordo che le persone che avete espulso dagli ammortizzatori sociali non potranno fare richiesta per il REI perché hanno nel 2016

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, come sappiamo, la nota di aggiornamento al DEF 2017,

sostiene questo quadro con una revisione al rialzo delle stime tendenziali sull'andamento dell'economia italiana rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, per tutto il quadriennio 2017- 2020, e in particolare per l'anno in corso che stima la crescita all'1,5 Tuttavia queste indicazioni favorevoli, a nostro avviso, non dovrebbero indurre il Governo nell'errore di ritenere che nella seconda parte del 2017 l'espansione economica continui quantomeno in linea con il ritmo del primo semestre, trainata dal settore manifatturiero e da alcuni comparti dei servizi, proprio in virtù del fatto che quelli citati a supporto di questa previsione sono indicatori congiunturali, vale a dire che siamo di fronte a dati di crescita non già strutturale, bensì solo indotta. Attenzione allora a dare per acquisiti obiettivi che sono ben lontani dall'essere raggiunti e consolidati. La storica divergenza del Paese, inoltre, nei tassi di crescita rispetto alla media europea suggerirebbe una cautela ulteriore. Questa cautela trova un'ampia e documentata conferma nell'andamento delle importazioni

Vorrei soffermarmi ora sul mercato del lavoro. Nella nota il tasso di occupazione è previsto superare il 58 per cento già nel 2017, per raggiungere il traguardo del 60 per cento In questo contesto, superata la fase critica del mercato del lavoro occorre secondo noi intervenire per rendere stabili i miglioramenti e avviare concretamente politiche del lavoro in grado di far aumentare i salari e ridurre i costi per le imprese. In altri termini, occorre attivare misure in grado di ridurre le tasse sul lavoro, non il contrario, come invece sento dire in questi giorni da autorevoli voci della sinistra. Mi riferisco al possibile, ennesimo rincaro delle tasse sul lavoro per compensare la *performance* deludente del *jobs act*. L'idea di usare la leva fiscale, aumentando il prelievo contributivo per scoraggiare i contratti a termine in favore di quelli a tempo indeterminato, non a caso raccoglie consensi in gran parte del fronte sindacale. Lo stesso presidente della BCE qualche giorno fa è tornato a incoraggiare i Governi a superare la politica dei *bonus* per concentrarsi piuttosto sul creare occasioni di lavoro, e non a caso ha citato tra i Paesi più indietro proprio l'Italia, il cui tasso di disoccupazione per gli *under* 25 a luglio era addirittura al 35,5 Ebbene, finché il Governo continuerà a muoversi in questa logica, senza affrontare le vere esigenze delle imprese italiane, in termini di competitività, innovazione e mercato, non si avrà mai un vero rilancio dell'occupazione, che sia stabile e duraturo. del fatto che questa politica suona come una beffa per tutti quegli imprenditori e - vi assicuro - e sono tanti che, nonostante questi anni di crisi, sono riusciti a non licenziare nessuno. Qual è il messaggio per loro? Volete accedere agli aiuti del Governo? Fatevi furbi. Licenziate per poi riassumere. Anche per questo, invitiamo il Governo a far propria la nostra proposta, inserendola nella legge di stabilità. Perché su questo punto occorre invece promuovere misure di riduzione del carico fiscale alle imprese che sia calcolato non sui nuovi assunti, che in questi anni hanno ingenerato meccanismi inefficienti, ma calibrata sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato e, soprattutto, che premiano le aziende che in questi anni di recessione hanno continuato a garantire il lavoro. La misura dello sgravio deve riguardare tutti i lavoratori e, quindi, anche i giovani. Una misura che quindi non deve rappresentare una discriminazione ma un principio di equità. Anche su questo punto non possiamo essere d'accordo. La manovra dovrà aggredire le inefficienze della spesa e non potrà ancora una volta tartassare i contribuenti. Perché il rischio più concreto è che una manovra troppo spinta verso le entrate possa bloccare i timidi segnali di crescita e sprofondare nuovamente il Paese nella recessione. Anche su questo punto, invece, la Nota dell'Esecutivo tradisce totale mancanza di coraggio politico e di visione strategica.

ho accolto con favore gli annunci del ministro De Vincenti per l'elaborazione all'interno della legge di stabilità, di una strategia possibile su zone economiche speciali, peraltro ancora tutte da definire. Però, rilevo che mentre nella scorsa legge di stabilità lo sgravio per le nuove assunzioni dei giovani al Sud era del 100 per cento, oggi il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale tale sgravio - il che ci soddisfa - ma lo ha ridotto al 50

Signor Presidente, questa cornice alla prossima manovra finanziaria, alla prossima legge di bilancio, è una cornice ottimistica. Tonino Guerra diceva che l'ottimismo è il sale della vita. Tuttavia, mi sembra che qui ci sia stato un eccesso di ottimismo perché, sì, il quadro economico internazionale migliora, tutti corrono ma noi corriamo meno degli altri. È lo stesso Governo a dire che nei prossimi tre anni l'esportazione calerà. Quindi, rifare tutta la crescita del PIL sull'immobiliare in ripresa e sui macchinari che vengono rinnovati sembra ottimistico (troppo) e, quindi, anche il discorso di mantenere l'inflazione al 2 con il *quantitative easing* ha fatto un miracolo, ma i miracoli non possono diventare strutturali. L'aumento dell'inflazione, quindi, appare non possibile con questi numeri.

e far ripartire sul serio l'economia ricorrendo a spese in *deficit* e a un contemporaneo aumento della pressione fiscale. È lo stesso Ufficio parlamentare del bilancio che pone dubbi e ci invita a rivedere al ribasso i dati forniti.

non aumentano, nonostante l'estrema necessità. La stessa Corte dei conti ci avverte dicendo che ciò può portare a ulteriori ferite nell'animo dei malati. I LEA rischiano di trasformarsi in un miraggio. Un motto popolare recita: «Chi è sano non sa quanto sia ricco». Auguro quindi a tutti gli italiani di rimanere in buona salute, perché lo Stato e la classe politica che ci dirige appaiono se non malati, almeno poveri. alla povertà di visione politica, di coraggio, di lungimiranza, di senso di giustizia, Povera di pietas! Eppure io spero, spero ancora che ci sia in Parlamento, in occasione dell'approvazione della prossima legge di bilancio, la maggioranza tra noi che possa e voglia avere uno moto di umanità moto di umanità e ricordare che non si possono separare i problemi sociali da quelli sanitari per tornare a comportarci, in scienza e coscienza, a vantaggio del bene di chi ne ha più bisogno: i malati. **Testo

condivido la Nota di aggiornamento al DEF nell'impostazione del Governo per gli obiettivi che vengono fissati e sottoscrivo gli interventi svolti dai colleghi Guerrieri Paleotti, Zanoni e Bianco. Mi limiterò quindi a fissare alcuni punti che credo il Governo debba valutare in maniera più approfondita. Oggi abbiamo un'emergenza dal punto di vista dell'occupazione, che riguarda in particolare i giovani. Il Governo ha giustamente fissato nell'occupazione giovanile una delle priorità. Credo però che il volume della disoccupazione giovanile al 35 per cento, rispetto a quella generale che si attesta all'11 del livello del problema e dell'emergenza, unitamente alla forte migrazione di giovani dal nostro Paese. Credo che il Governo debba compiere uno sforzo per recuperare risorse aggiuntive e aggredire in maniera più forte il problema della disoccupazione giovanile. Signor Ministro, nella Nota di aggiornamento al DEF avete fatto una valutazione, ma vorrei che almeno qualcuno del Governo mi ascoltasse, perché vi vedo tutti impegnati in altre conversazioni.

e giustamente avete dato conto di una sostenibilità del debito pubblico e della capacità del nostro Paese di reggere anche a uno *choc* che possa derivare da tensioni geopolitiche o da altri elementi.

di investimenti pubblici in infrastrutture. Anche il risultato importante del venir meno del Patto di stabilità non ha fatto crescere gli investimenti nei Comuni. Per un comparto importante della nostra economia come le costruzioni siamo solo all'inizio di una ripresa. Accanto al tema dello sviluppo del Sud, quindi, abbiamo un bacino di potenzialità enormi su cui crescere. Tuttavia le infrastrutture e gli investimenti pubblici continuano a tardare,

Medioriente. Attraverso l'allargamento del Canale di Suez del 2015, il volume dei traffici a Suez è quattro volte quello del Canale di Panama. Questo

all'area dell'Africa, al Medioriente e al Nord Europa come *hub* per i traffici per la sponda atlantica degli USA - ha rimesso il Mediterraneo davvero al centro del commercio internazionale. È lo snodo strategico. Pertanto, tutti gli investimenti in infrastrutture e logistica per il Centro-Sud rappresentano un

una ripresa strutturale del nostro Paese e porlo alla testa dell'Europa, mancando ancora tutta la componente investimenti pubblici in infrastrutture, con questa opportunità credo che il nostro Paese abbia davanti una prospettiva straordinaria.

sia possibile essere così sfacciatamente ottimisti sull'andamento economico del nostro Paese. Ci chiediamo ancora una volta in che mondo viviate: per una volta tanto, ahimè, sono d'accordo con il collega Brunetta. Signor

coloro che si lamentano e che non vedono una prospettiva per il loro futuro? Incontro solo io i giovani che stanno facendo la valigetta perché se ne stanno andando da questo Paese? Sono giovani che abbiamo formato, su cui giustamente

D'altronde, voi siete il clone del Governo Renzi. I Governi che si stanno succedendo sono quelli dei proclami e degli annunci, ma nei fatti concreti - ahimè - state

l'infrastruttura Rotterdam-Genova. Con il raddoppio del Canale di Suez, la piattaforma del nostro Paese nell'ambito delle infrastrutture potrà essere

Vi esorto a lasciar stare in questo momento la possibile fusione tra Ferrovie e ANAS; non sommate a casino altro casino. Cerchiamo di terminare questa legislatura; chiudete i conti "alla bell'e meglio".

vi manderanno a casa e speriamo che chi verrà dopo di voi abbia almeno il pudore di non fare strane alchimie dal punto di vista economico e di raccontare la realtà di un Paese che fa grande

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Nota di aggiornamento del DEF, che stiamo discutendo, dovrebbe certificare un dato importantissimo, ossia il calo del debito pubblico dello 0,1-0,2 per cento a partire dal 2017. È quindi necessario evidenziare che si tratta di un'inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi dieci anni. Certo, lo *slogan* "più PIL, meno debito" con cui il Governo ha presentato la Nota va riempito coerentemente di contenuti nella prossima manovra economica, ma, in effetti, rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile (+1,2 per cento), la variazione reale del PIL, a fine 2017, dovrebbe essere pari +1,5 rispetto all'anno precedente e la stessa crescita dovrebbe ripetersi nel 2018 e nel 2019, il che significa che il tasso di crescita del PIL è stato rivisto al rialzo di circa il 25 per cento in termini relativi. Va vista in positivo anche la rinuncia alle clausole di salvaguardia, dato che il mancato gettito di circa 15 miliardi di euro di IVA si tradurrà in circa 5 miliardi di euro in più di produzione e reddito, trainati dai maggiori consumi. Crescerà lievemente il *deficit*, ma il rapporto tra *defìcit* e PIL per il 2018, previsto pari all'1,6 per cento contro l'1,2 per cento indicato ad aprile, resta pur sempre molto al di sotto del limite del 3 In definitiva, si va verso una maggiore crescita del PIL nominale, un maggior contenimento del fabbisogno della pubblica amministrazione e un maggior ricorso alle privatizzazioni, il cui introito andrà ad abbattere lo *stock* del debito. Queste sono le premesse sostanziali e oggettive che noi colleghi del Gruppo ALA-Scelta Civica abbiamo preso in considerazione, analizzando i dati e approcciandoci al testo con lo spirito costruttivo e riformista che da sempre ha caratterizzato le nostre scelte parlamentari. Fatte queste premesse, è importante ricordare che in questi mesi non abbiamo votato la fiducia al Governo Gentiloni ma che sui provvedimenti utili al Paese non abbiamo mai fatto mancare il nostro apporto, pur se talvolta critico. Anche in questo caso, pur essendo critici ci siamo soffermati sulla necessità e sulle prospettive che la Nota di aggiornamento al DEF può portare. Di certo il testo può essere definito equilibrato e in linea con la timida ripresa economica che va consolidata. Inoltre, l'approccio costruttivo con cui voteremo questo DEF è dato anche dalla convinzione che un voto non risicato del Parlamento possa dare al Governo più forza quando dovrà trattare con la Commissione europea. Quando un Presidente del Consiglio del nostro Paese tratta con l'Europa per cercare di portare più Italia e un'Italia più forte nell'Unione europea, quello è sempre il nostro Presidente del Consiglio. Nessuno che abbia un briciolo di responsabilità politica può augurarsi l'arrivo della *trojka*, ma neppure un DEF tutto orientato ai canoni della vecchia sinistra "tassa e spendi".

le ragioni che lo portano ad ignorarli. Il primo tema riguarda il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL. La Nota di aggiornamento del DEF si limita ad osservare che, siccome il PIL cresce e la spesa viene mantenuta allo stesso livello che era stato indicato quando non avevamo ancora

Quello che sentenzia la Nota di aggiornamento del DEF è che, non solo non si avvia un percorso di riallineamento, ma si aumenta la caduta di questo rapporto e certamente, in un momento in cui il PIL aumenta, ci si sarebbe aspettati che fosse prestata attenzione anche ad un'adeguata, perlomeno analoga, crescita della spesa sanitaria. Questo - mi dispiace dirlo - non fa che confermare quanto abbiamo tante volte lamentato e cioè che la politica per la salute non è nell'agenda del Governo e che si continua quindi a considerare la politica della salute come quella in cui si possono aumentare le restrizioni, anziché aiutare il sistema a migliorare il proprio funzionamento. Dico per inciso - molto è già stato detto da chi mi ha preceduto che negli ultimi cinque anni la sanità, che è un settore ad alta intensità di lavoro, ha perso quasi 40.000 dipendenti e, siccome è un settore ad alta intensità di lavoro e non può produrre prestazioni se non ha i lavoratori, ricorre ovviamente all'*outsourcing*, a forme di somministrazione del lavoro che costano molto di più di quanto non costerebbe assumere dipendenti. Un secondo tema tema riguarda la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa e delle esenzioni. Anche questo è un impegno che nel 2014 il Governo si è assunto con il Patto per la salute, in cui, all'articolo 8, è scritto che, a partire dalla costituzione di un gruppo di lavoro, si sarebbe rivisto

e produce effetti di iniquità sempre più gravosi in una situazione difficile come quella in cui si trovano tanti milioni di cittadini italiani. Su questo penso che sia necessario cominciare a dare un segnale, perché altrimenti non si può che concludere, in modo imbarazzante, che la disattenzione nei confronti della sanità pubblica non è dovuta alla crisi, ma ad una scelta esplicita del Governo. Signor Presidente, colleghi, negli ultimi tempi abbiamo ascoltato, sul fronte economico, buone notizie, ora confermate da questa Nota di aggiornamento: la ripresa economica si è consolidata negli ultimi mesi con una crescita del PIL dell'1,5 per cento, invece del previsto 1,1 per cento della previsione di aprile scorso. La disoccupazione è in calo, mentre aumenta l'occupazione. In questo scenario positivo mi soffermo su un punto che ritengo particolarmente importante, ovvero la necessità di uno sviluppo ambientalmente sostenibile. Mi auguro vivamente che la ripresa a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e che si sta consolidando negli ultimi mesi si discosti dalle esperienze precedenti, nelle quali, alla crescita economica, sono spesso corrisposti fenomeni ambientalmente negativi. Mi riferisco, ad esempio, a una crescita delle emissioni di CO2 direttamente proporzionale a un incremento del PIL o a un aumento della produzione di rifiuti *pro capite*, anch'esso associato alla crescita economica. E questi sono solo alcuni esempi. Questo non deve più avvenire, non solo per i danni che porterebbe all'ambiente in cui viviamo, Grazie a tutta la citazione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e quelli ambientalmente favorevoli come strumento conoscitivo per favorire una transizione verso un sistema fiscale ecologico. Ricordo che i SAD rappresentano oltre 16 miliardi di euro, mentre i SAF superano di poco i 15,5 miliardi di euro. Sono maggiori i sussidi dannosi all'ambiente rispetto a quelli favorevoli. Se si potesse, con un colpo di bacchetta magica, eliminare i sussidi dannosi all'ambiente non solo si farebbe un grande favore all'ambiente ma si recupererebbero oltre 16 miliardi. Su questo occorre quindi intervenire. Nel predetto catalogo, predetto catalogo, prodotto dal Ministero dell'ambiente come prescritto dall'articolo 68 del collegato ambientale del 2015, vi sono anche riportati le raccomandazioni e i suggerimenti proposti da vari organismi internazionali, fra i quali l'Agenzia europea per l'ambiente, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il Parlamento europeo. Le proposte per intervenire sulle politiche fiscali ambientali quindi non mancano. Non occorre avere molta fantasia e non ritengo necessaria l'istituzione di alcuna Commissione dedicata, come fu in passato, ad esempio, la Commissione Marè che, tra l'altro, non aveva alcun membro del Ministero dell'ambiente. Mi aspetto che, in quest'ottica, la futura legge di bilancio intraprenda un percorso di riduzione dei SAD (sussidi ambientalmente dannosi) e magari anche un incremento di quelli ambientalmente favorevoli. Non resti solo una semplice citazione nella Nota, ma si concretizzi con concreti ed efficaci interventi. Il sistema fiscale può e deve essere strumento di una politica economica sostenibile, se riduce alcuni sussidi che non solo talvolta distorcono il mercato, ma sostengono pratiche ambientalmente dannose. Una delle raccomandazioni della Commissione europea, citata nella Nota del DEF, indica proprio cito testualmente - «un'azione decisa per ridurre il numero e l'entità delle agevolazioni fiscali». È una affermazione che non mi convince in valore assoluto, ma è sicuramente auspicabile per i sussidi ambientalmente dannosi. Oltre all'intervento fiscale bisogna potenziare tutte le occasioni e le situazioni per le quali i cittadini e le aziende intraprendano azioni ambientalmente virtuose. Ad esempio, Ad esempio, è stato recentemente introdotto, da una direttiva europea, l'obbligo per le aziende con oltre 500 dipendenti e con un certo fatturato di una relazione non-finanziaria che indichi l'impatto sociale e ambientale delle attività dell'azienda È un modo, ancora troppo timido e limitato dal mio punto di vista, di incrementare e valorizzare la responsabilità sociale e ambientale delle aziende. Occorre spingersi oltre in questa direzione prevedendo, ad esempio, adeguata pubblicità alle dichiarazioni delle aziende in questa relazione. Come sappiamo, le aziende sono sempre più attente alla reputazione e all'immagine che hanno presso il pubblico. Un'azienda che dichiarasse un forte impatto negativo sull'ambiente, ad esempio, avrebbe un conseguente impatto negativo sul proprio fatturato per la reazione negativa della sua clientela. Non è un processo rapido di crescita della consapevolezza degli impatti, ma su questo occorre intervenire, magari sanzionando fortemente le dichiarazioni mendaci che si trovassero in queste relazioni non-finanziarie e rendendone adeguata pubblicità. PRESIDENTE. È iscritta

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016, del 2016, in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati del prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione

il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8

di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento di oggi. Un altro fattore determinante dell'attuale congiuntura favorevole è l'effetto cumulato delle riforme strutturali intraprese negli ultimi anni, da quella della pubblica amministrazione, a quella del mercato del lavoro, a quella della finanza per la crescita, fino ad arrivare a quelle relative all'efficienza del fisco e alla giustizia. e alla giustizia. Nello scorso mese di agosto, per la prima volta in Italia, è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che introduce significative novità in tema di servizi finanziari, assicurativi e professionali, mercato dell'energia, l'obiettivo del provvedimento è di rilanciare la modernizzazione dei comparti coinvolti, stimolare la produttività e la crescita, consentendo ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a costi inferiori. Questo scenario non nasce dal nulla ma è frutto di oltre quattro anni di scelte politiche mirate e lungimiranti che ci permettono, oggi, sulla base dei segnali incoraggianti degli anni scorsi, di affrontare il futuro non più col semplice ottimismo

a investitori italiani ed esteri di settori quali le farmacie e gli studi legali, un punto, questo, sul quale Alternativa popolare si è battuta strenuamente durante questi anni al governo, riuscendo ad indirizzare, molto spesso in maniera determinante, le politiche del governo nel settore delle professioni, riuscendo così, finalmente, ad indurre i nostri *partner* di governo a superare quella diffidenza verso questo questo molto che è costata al Paese e a un settore fondamentale del nostro Pil un ingiustificabile ritardo. Un'ulteriore spinta all'economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. Il Governo è da tempo all'opera per promuovere un'inversione di tendenza degli investimenti pubblici. Ciò affinché venga non solo stimolata la domanda aggregata, ma migliori anche il potenziale di crescita dell'economia attraverso infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili, Anche su questo tema, inutile ricordarlo, la nostra cultura liberale, contraria ad investimenti pubblici a pioggia e senza alcun criterio, ha evitato il ripetersi dello sperpero di risorse pubbliche messo in atto negli anni passati. Nonostante il periodo post-crisi, grazie ad un intelligente ri-allocamento delle risorse destinate alla crescita, siamo riusciti ad portare avanti un piano di investimenti pubblici mirati e sulla base delle reali esigenze dei settori e dei territori ai quali sono rivolti. Le relative clausole di salvaguardia sono state modificate con la manovra di primavera, riducendone l'importo rispetto alla Legge di Bilancio 2017 in misura che varia fra 3,8 miliardi nel 2018 e 4,4 miliardi nel 2019. L'impatto negativo sul PIL è quindi lievemente inferiore rispetto alle previsioni di aprile, soprattutto nel 2018. La nuova previsione tendenziale del PIL per il 2018 riflette anche il maggior effetto di trascinamento derivante dalla revisione al rialzo del profilo trimestrale di crescita reale durante il 2017, il quale vale circa 0,1 punti percentuali di crescita. Chiaramente l'azione del Governo e della maggioranza sarà rivolta alla disattivazione delle suddette clausole relativamente all'anno 2018. Nel primo semestre dell'anno, in coerenza con il quadro programmatico di finanza pubblica del DEF 2017, il Governo ha adottato alcuni provvedimenti con carattere di urgenza che associano misure di consolidamento degli andamenti di finanza pubblica a interventi per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nonché iniziative per gli Enti territoriali, per il rilancio della crescita economica nel Mezzogiorno e per la gestione del fenomeno migratorio.

recate dal decreto legislativo n. 50 del 2017, per l'anno 2017, il miglioramento del saldo strutturale di bilancio risulta pari a circa lo (3,4 miliardi). Negli anni successivi sono attesi lievi effetti migliorativi per tutti i saldi di finanza pubblica. Le risorse reperite in termini di manovra lorda ammontano a 5,2 miliardi nel 2017, aumentano a 10,2

per circa 2,62 miliardi, attestandosi per la prima volta a 14,1 miliardi di euro. Si tratta, in particolare, dell'estensione del meccanismo dello *split payment* a tutta la pubblica amministrazione, ai professionisti, amministrazione centrale e locale nonché alle società quotate in borsa, e delle disposizioni che mirano a limitare gli abusi dell'istituto delle compensazioni fiscali. il patrimonio immobiliare, il piano di valorizzazione del Governo si sviluppa secondo due principali direttrici: la messa a reddito dei cespiti più appetibili, attraverso variazioni nella destinazione d'uso degli immobili, il loro conferimento a fondi di gestione del risparmio per la successiva In conclusione, sono risultati che incoraggiano a proseguire il percorso intrapreso per rafforzare ulteriormente una ripresa dell'economia italiana che, dopo anni di profonda recessione, si è manifestata nel 2014, nel 2014, consolidata nel biennio 2015-2016 ed ha, infine, preso vigore nell'anno in corso, anche in virtù di un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, mostrando soprattutto crescenti segnali di irrobustimento strutturale. Su questi e su molti altri obiettivi centrati Alternativa Popolare ha investito tutte le proprie energie, garantendo a questo Governo una maggioranza stabile, in grado di porre in essere tutti quei provvedimenti normativi che, a più di quattro anni di distanza dall'aprile 2013, consegnano agli italiani un quadro sensibilmente migliorato La crescita del prodotto interno lordo negli ultimi trimestri ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi turistici hanno accelerato e c'è stata una graduale ripresa degli investimenti. Tutto ciò fornisce, nel complesso, segnali incoraggianti, particolarmente evidenti nella recente La principale sfida per la politica economica è trasformare l'attuale fase di uscita dalla crisi in una ripresa robusta e strutturale, che permetta all'Italia di superare definitivamente una prolungata stagione caratterizzata dal ristagno della produttività e della crescita. Il percorso da compiere è ancora lungo, benché alcune riforme comincino a produrre effetti concreti. in nome di una stabilità che dovrebbe essere garantita ad ogni Paese e per ogni Governo. Le famiglie, le imprese e i lavoratori oggi, grazie a questo intenso e complesso lavoro, possono guardare il passato come un lontano ricordo. L'Italia è ripartita e cresce di nuovo, nonostante le enormi difficoltà che in partenza potevano far temere il contrario. Grazie a tutta questa lunga serie di riforme e di investimenti ci apprestiamo a consegnare al prossimo Parlamento un'Italia non solo più stabile e più florida, ma con reali prospettive di miglioramento. Una sfida che sembrava impossibile e che pure siamo riusciti a vincere, superando le storiche contrapposizioni ideologiche che per anni hanno ingessato la nostra economia a schemi ormai, finalmente, davvero superati. Signor Presidente, Presidente, utilizzerò questi minuti per annunciare quale sarà il voto Grazie Grazie

Sullo scostamento abbiamo avuto sempre una posizione chiara, critica del contenuto dell'articolo 81 della Costituzione (così com'è stato novellato, con l'obbligo di pareggio di bilancio), perché abbiamo sempre pensato che l'indebitamento sia uno strumento che deve rimanere nelle mani del Parlamento, per decidere quale tipo di promozione e di sostegno all'economia sia utile (ogni esercizio, in ogni circostanza). L'altra questione riguarda la decisione del voto sulla Nota di aggiornamento. Siamo alla vigilia - è evidente - di una campagna elettorale e la Nota di aggiornamento che è stata presentata dal Governo ha numeri più confortanti di altri che abbiamo visto in questa legislatura. Per questa ragione, per l'uso che si fa di una parte delle dotazioni finanziarie che la crescita registrata negli ultimi dieci trimestri in modo costante garantisce, per l'impegno verso lo stato sociale e verso misure di contrasto alla povertà che è stato assunto e pubblicamente dichiarato dal presidente Gentiloni Silveri, per noi merita questo atto di fiducia. Poi vedremo la manovra di bilancio, vedremo le cifre e vedremo come verranno orientate. Mi permetto, signor Presidente, di fare una valutazione di tipo politico

La valutazione di tipo politico è la seguente. Noi viviamo un momento tormentato, lo viviamo nel nostro continente, lo viviamo all'interno dell'eurozona, lo viviamo soprattutto nel Mediterraneo. E non sono solo i flussi migratori il tema, ma sono soprattutto le ragioni dei flussi migratori che noi dobbiamo affrontare in queste settimane, in questi mesi e in questi anni, cioè un Mediterraneo sconvolto sistematicamente da decenni di guerre, da un'aggressione ormai insopportabile delle antiche civiltà del bacino del Mediterraneo nel suo complesso, dal Medio Oriente al Nord Africa, alle pendici della nostra Europa.

voglio concludere dicendo che forse bisogna anche rivalutare la funzione della politica, riconoscendo a ciascuno di noi un tratto di buona fede ed evitando i giudizi personali sulle posizioni politiche. Mi rivolgo anche ai compagni di MDP e ai miei stessi compagni di Campo progressista, perché questo Gruppo è mio patrimonio esattamente come di tutti gli altri che lo compongono. come di tutti gli altri che lo compongono. È patrimonio mio, del sindaco della mia città, Massimo Zedda, e di tutti coloro che hanno contribuito quotidianamente a dare un segnale politico nuovo verso un centro-sinistra e un'area democratica in pieno sviluppo, così da fornire al Paese un'occasione vera di rilancio della nostra economia e della nostra società. Non saremo mai strumentali, mai strumentali, ma assolutamente più che sensibili ai diritti di tutti gli altri a manifestare le loro opinioni politiche e le loro posizioni. Noi rispettiamo le posizioni degli altri perché è giusto, questo è il Parlamento ed è giusto che tutti noi ne abbiamo diverse e noi le mettiamo a confronto senza mai colpire coloro che se ne fanno carico, ma anzi aiutandoli ad esprimere liberamente il loro pensiero. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anche questo secondo documento previsionale del Governo Gentiloni Silveri conferma la *ratio* della politica economica dei Governi di centro-sinistra dal 2014 ad oggi. Con l'intento di fare crescita è stata utilizzata soprattutto la leva del *deficit* di bilancio. L'effetto espansivo sul PIL si è però rivelato quantitativamente inferiore a quanto raccolto in più sul mercato finanziario. Per capirci con qualche semplice numero: dopo quattro anni e oltre 164 miliardi di spesa in *deficit* abbiamo un PIL a 1.716,5 miliardi, cioè 26 miliardi in meno di quanto atteso nel 2014. Tutti i documenti programmatici, e le relative manovre, hanno via via posticipato l'obiettivo del pareggio di bilancio che, inizialmente previsto per il 2018, viene ora rinviato al 2021. E il maggior *deficit* per il prossimo anno (0,6 in più sul tendenziale), in realtà è di 1,9 punti percentuali maggiore rispetto al dato previsionale del primo DEF Buona parte del maggiore indebitamento netto verrà utilizzato per coprire le clausola di salvaguardia per il 2018, scongiurando il previsto aumento delle aliquote IVA all'11,5 e al 25 per cento, e una parte dell'aumento per il 2019. E, quindi, rimangono ulteriori 45 miliardi di clausole dal 2019 al 2021, che dovranno essere disinnescate dal prossimo Governo. Guardando la tabella allegata all'audizione di ieri del Ministro

- vale lo 0,31. Cioè tutte le altre misure, lodate e decantate, avranno un impatto dello 0,01 del PIL. Si avranno nuove entrate per 5,1 miliardi e ciò significa: nuovi condoni fiscali, nuove tasse ovvero riduzione di agevolazioni fiscali, cioè, comunque tasse che si abbatteranno su professionisti, su lavoratori e su lavoratori autonomi. Lo *stock* del debito, intanto, è salito oltre i 2.300 miliardi, grazie a una spesa pubblica cresciuta senza sosta. Riassumendo qualche dato, dal 2014 al 2017 si sono avuti 156 miliardi di maggiore PIL, 164 miliardi di maggiore spesa in *deficit* e 233 miliardi aggiunti allo *stock* del debito. Questi dati sconfessano i partigiani della spesa a ogni costo. La spesa deve essere di qualità

Si tratta di risorse vere tolte agli investimenti. Non basta, quindi, la riduzione del rapporto debito/PIL: è necessaria una riduzione dello *stock* prima che risalgano gli oneri per farvi fronte.

al conto consolidato dello Stato, per liberare risorse per gli investimenti. A questo va aggiunto un responsabile intervento sulle società partecipate, per le quali le cosiddette riforme di questa legislatura si stanno rivelando assolutamente inadeguate. E preso atto che sono previsti circa 500.000 esodi dalla PA verso gli enti di previdenza pubblica, prima di ogni *turnover* su piante organiche ormai obsolete, andranno verificate le effettive necessità del perimetro pubblico, che conta un lavoratore su sette in Italia. Ugualmente bisognerà eseguire interventi per rendere dinamico e inclusivo il mercato del lavoro, regolato ormai dalla legge Fornero, che impedisce agli ultracinquantenni di andare in pensione

la NADEF programma i conti pubblici non su interventi strutturali, ma ancora sulle variabili esogene, che vedono l'economia del mondo in un ciclo favorevole di crescita. Le riforme credibili sono mancate negli ultimi quattro anni caratterizzati da *bonus* in uscita, *una tantum* in entrata e una spesa pubblica improduttiva in crescita, al posto di una oculata *spending La fuga degli investimenti dal nostro Paese - pari a una cifra che è quasi un decimo del PIL italiano - è, purtroppo, il giudizio più obiettivo e più severo che viene dato all'azione dei Governi di centro-sinistra. Si tratta di somme che torneranno in Italia per innescare una crescita permanente dell'economia, quando ci saranno politiche di Governo autorevoli e riforme autentiche.

Signor Presidente, Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi, la Nota di aggiornamento del DEF

la crescita riducendo - questo mi pare il dato rilevante - notevolmente il differenziale con il ritmo degli altri Paesi europei. Sono molto positivi i dati sull'occupazione che, mese per mese, migliorano, riducendo soprattutto la piaga della disoccupazione e rilevando anche qualche positività su quella giovanile.

il sostegno agli investimenti pubblici e privati, un forte impulso all'occupazione giovanile e una rilevante politica di carattere sociale che si pone in questo momento come necessità rispetto alle gravi ferite che la crisi degli ultimi anni ha lasciato Su economia e lavoro vanno valorizzati tutti gli elementi, in particolare quelli di forte legame con l'innovazione e la qualità, che diano più forza e più respiro alle prospettive di crescita. Il tema dell'impresa 4.0, con investimenti in tecnologia digitale fortemente incentivati, va - a mio avviso - collegato ad altri fattori per renderlo completo. E mi riferisco, innanzitutto, al completamento rapido del programma di investimenti nel territorio della banda ultralarga - l'Italia su questo è ancora, purtroppo, molto diseguale tra grandi centri, aree interne e territori più marginali - in tempi più solleciti di quanto sta avvenendo;

delle modalità diverse di pagamento dell'IVA della fatturazione elettronica, ci troviamo a impattare pesantemente con le difficoltà nella pubblica amministrazione. Quindi, se vogliamo che gli investimenti abbiano un effetto moltiplicatore, bisogna agire anche più rapidamente sulla trasformazione dell'economia digitale. Sul piano degli investimenti, vanno fortemente spinti gli investimenti pubblici, sia attuando con le cadenze previste il programma molto positivo del Fondo investimenti, varato nel mese di luglio; sia rafforzando - e questo è un punto delicato, in quanto sono necessarie risorse - la possibilità di investimento degli enti locali, allargando la possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che in molte realtà è presente - e potrebbe diventare immediatamente investimento nell'ambito - per esempio - o nei lavori legati agli enti locali - ma purtroppo, pur nello sblocco del Patto di stabilità, risente ancora dei limiti che conosciamo. Oltre a questo, bisogna lavorare molto fortemente sul tema dell'occupazione. È molto positivo il dato dell'incremento o, meglio, della riduzione della contribuzione per favorire l'occupazione giovanile. È molto importante collegare, anche sul piano dell'occupazione, il tema della trasformazione industriale. Quindi, accanto a impresa 4.0 bisogna pensare anche alle prospettive di un lavoro 4.0, con gli adeguati sostegni all'attività permanente di formazione. Infine, la seconda gamba è il tema delle politiche di carattere sociale. Segnalo tre argomenti su questo punto ai quali prestare molta attenzione. come prevede anche la Nota di aggiornamento nella tabella che abbiamo esaminato ieri - riguarda il rafforzamento per quanto riguarda il reddito di inclusione. È una misura importante, andrà in vigore dal primo gennaio razionalizzando le sperimentazioni esistenti, che deve immediatamente entrare in rapporto con la realtà della sofferenza sociale attraverso misure concrete e, quindi, avrà bisogno di essere ulteriormente rafforzata sul piano dell'investimento. È importante - come hanno già detto altri - valutare l'impatto delle misure di risparmio nel mondo sanitario con le condizioni reali

le gravi problematiche che ancora insistono, soprattutto quando un lavoratore in età avanzata fa lavori molto pesanti perde il lavoro per la crisi.

Tenere insieme crescita, sviluppo e occupazione vuol dire prestare grande attenzione alla solidarietà sociale e alle politiche sociali. è pervenuta alla Presidenza, sulla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, la proposta di risoluzione n. 100, dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller. Sono inoltre pervenute alla Presidenza, sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017, le seguenti proposte di risoluzione:

limiterò a una breve replica, perché il dibattito che è seguito mi sembra abbia toccato molti punti

l'economia italiana è tornata su un sentiero di crescita relativamente elevato. all'interno di un processo di aggiustamento che sta in qualche modo garantendo un consolidamento dei nostri conti pubblici. Il dato più importante è che si profila una compatibilità tra questi due obiettivi, e quindi la possibilità di allargare lo spazio di crescita che si apre in prospettiva. Certamente la fase è stata molto favorevole, un'occasione positiva data da un contesto europeo e internazionale che ha favorito il processo di aggiustamento. Ma non ci sono dubbi che una tale opportunità sia stata sia stata colta al meglio attraverso misure e politiche che non hanno solo guardato al breve periodo, ma hanno anche considerato obiettivi di medio e lungo termine. Come ho sottolineato nella parte finale della mia

l'obiettivo di colmare quella distanza che ancora oggi ci separa dalla media dell'area dell'euro è pienamente nelle potenzialità del nostro Paese; dall'altro, è allo stesso tempo nelle potenzialità del nostro Paese Paese cogliere le grandi opportunità date dalle trasformazioni in atto. Non dimentichiamo che si stanno aprendo nuovi orizzonti sul piano del rinnovamento dell'organizzazione della

di parlare il ministro dell'economia e delle finanze, professor Padoan, al quale chiedo di esprimere il parere sulla proposta di risoluzione presentata alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243

il Governo condivide la proposta di risoluzione n. 100, ai fini della relazione al Parlamento, a firma Zanda, Bianconi e Zeller. In secondo luogo, per quanto riguarda la Nota di aggiornamento al DEF, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 5 a firma Zanda, Bianconi e Zeller. Signor Presidente, farò alcune brevi considerazioni alla luce del dibattito che si è svolto. Innanzi tutto, è un dato di fatto - credo nessuno possa negarlo

che, in base agli indicatori più diversi, ma che si rafforzano a vicenda, il quadro dell'economia italiana sta decisamente migliorando: dal punto di vista della crescita e dell'occupazione, i numeri sono chiari e anche la qualità del lavoro è chiara; dal punto di vista della finanza pubblica, si sta gradualmente ma decisamente consolidando, e ciò, per un Paese ad alto debito, come il nostro, continuamente sottoposto al vaglio dei mercati, prima ancora che delle istituzioni internazionali, è un elemento fondamentale. si rafforza in quantità e in estensione per settori e Regioni del Paese e i rischi finanziari si allontanano dal punto di vista sia della gestione del debito pubblico che della riparazione profonda avvenuta e che continua ad avvenire nel sistema bancario,

sentiero che deve vedere la finanza pubblica impegnata a sostenere - in quantità e in qualità - la crescita e l'occupazione e allo stesso tempo accelerare il consolidamento. Siamo un Paese ad alto debito, ma da noi il debito ha cominciato a scendere, e questo è stato certificato dall'ISTAT per il 2015 pochi giorni fa; è previsto nella Nota di aggiornamento al DEF per il 2017: continuerà a scendere in misura e con velocità crescente negli anni prossimi, togliendo dal tavolo un fattore di rischio che molto spesso, in passato, ha minacciato la possibilità di fare politica economica nel nostro Paese e che adesso, invece, ci offre un grado di libertà. L'impostazione di finanza pubblica, dal punto di vista dei limiti che deve rispettare, parte da un valore concordato in sede europea, che peraltro deve essere

che riconosce un principio che la politica economica del Governo negli ultimi anni ha sempre affermato, e cioè la necessità di contemperare crescita e consolidamento. Quindi, l'aggiustamento dello 0,3 strutturale, che con i dati del PIL oggi disponibili equivale a 1,6 di indebitamento, va in quella direzione. Ma l'ottimismo che viene citato, e non vedo cosa ci sia di male - in fondo, in passato, siamo stati tacciati di essere ottimisti, ma alla luce dei risultati siamo stati pessimisti rispetto a quello che effettivamente si è verificato verificato - non deve essere una ragione per fermarsi: al contrario, deve essere una ragione per accelerare lo sviluppo e renderlo strutturale e robusto; approfittare del momento ciclico favorevole a livello europeo e globale per rendere questa crescita, che è ancora in parte ciclica, permanente e duratura, con tassi di crescita che già sono superiori a quelli che, ancora prima della crisi finanziaria, caratterizzavano l'economia italiana. La Nota di aggiornamento al DEF definisce attualmente un quadro di riferimento di crescita, di macroeconomia e di finanza pubblica, che andrà riempito con una definizione di misure specifiche in base alla legge di bilancio. Ma già nella Nota di aggiornamento al DEF si indicano alcuni ambiti di intervento che, date le risorse limitate - come è chiaro a tutti - permettono innanzitutto di rimuovere completamente le clausole di salvaguardia, scongiurando quindi aumenti di IVA che, altrimenti, costituirebbero un fattore di freno della crescita e, pertanto, pericolo per il consolidamento della crescita se non disattivate. Il primo elemento è, quindi, la disattivazione di dette clausole. Detto ciò, nell'ambito dei vincoli di aggiustamento di bilancio concordati a livello europeo rimangono risorse limitate, che possono però però essere estremamente utili in un contesto di continuazione della strategia; una strategia che non esiterei a definire di crescita inclusiva, quindi di crescita del prodotto, di composizione del prodotto, ma di risorse che permettono a chi è ancora ai margini della ripresa di essere incluso in modo più efficace. Mi riferisco evidentemente alla disoccupazione giovanile, che peraltro è diminuita in base agli ultimi dati, ma che è ancora decisamente troppo alta; mi riferisco a spese per il grado di benessere generale nel Paese. È stata citata da molti oratori la questione del sistema sanitario: questo è sicuramente un ambito nel quale andranno valutate misure di miglioramento e di efficientamento. Per concludere, la crescita di un Paese avanzato in Europa, come il nostro, non può non basarsi su una visione del futuro fondata sull'incentivazione alla produttività, sull'innovazione, sul piano Impresa 4.0, e quindi sulla possibilità di crescere a tassi molto più sostenuti e sostenibili che in passato, malgrado l'invecchiamento della popolazione e un ambiente demografico avverso. Questo non solo è possibile, ma si sta cominciando a realizzare. Non bisogna, quindi, fermarsi e accontentarsi di quello che osserviamo: bisogna definire un programma di crescita per gli anni a venire. *(Applausi

«Per il 2018 la politica di bilancio continuerà a inscriversi nella strategia che, a partire dal 2014, ha assicurato una costante riduzione del rapporto *deficit-*PIL, la stabilizzazione del debito nonché la sua riduzione. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo punta al conseguimento del sostanziale pareggio di bilancio nel 2020 e all'accelerazione della riduzione del rapporto debito-PIL».

"più PIL, meno debito". Compulsando i numeri ci si accorge che in effetti, secondo le stime del DEF, qualche «zero virgola» di PIL potrebbe essere recuperato e qualche «zero virgola» di debito potrebbe essere abbattuto. Ma la politica del sentiero stretto tracciata dal ministro Padoan appare tutt'altro che tranquilla. Se infatti proseguiamo nell'esame dei dati, ci imbattiamo nelle cifre riferite al *deficit*, che invece salgono dall'1,2 per Io non sono un esperto di economia, ma mi domando: come si può ridurre il debito pubblico aumentando il *deficit*? Non credo occorra essere esperti per sapere che aumentare il *deficit* proprio adesso, in un periodo di seppur timida crescita, è quanto quanto di più sconsigliabile. A Via XX Settembre, evidentemente, si ritiene invece che fare più *deficit* è sempre meglio che farne meno, a prescindere dal ciclo economico, senza curarsi del contesto e delle tendenze macroeconomiche europee e internazionali. Eppure la lezione del 2011 dovrebbe insegnarci che, a furia di fare politiche procicliche, ci si ritrova a non avere spazio fiscale e a dover applicare tagli severi nel mezzo di una recessione, e cioè proprio quando fa più male. Colleghi, debito e *deficit* non sono e non potranno mai essere variabili scollegate. Il debito non è altro che la somma del *deficit* che si accumula anno dopo anno: il *deficit* di ieri è il debito di oggi; il *deficit* che ci proponete di aumentare oggi sarà il debito dei nostri figli. Non è tutto: la Nota di cui discutiamo è stata presentata basando il ragionamento su affermazioni puramente algebriche. Ma, se andiamo un po' più a fondo sulla natura dei dati, ci accorgiamo che lo stimato aumento del PIL non è dovuto a una ripresa stabile dei consumi, della produzione industriale, dei posti di lavoro, ma è invece, sostanzialmente, il risultato di una contromanovra. La lievissima previsione di rialzo del PIL non fotografa un'economia che cresce: si fonda piuttosto su una presunzione derivante dalla retromarcia sulle clausole di salvaguardia, che il Governo stesso aveva imposto, il cui mancato gettito non verrà recuperato con un piano serio di razionalizzazione della spesa, bensì con altro *deficit* e con generici tagli e aumenti di entrate, di cui non è dato conoscere il fondamento. Se il *trend* dei tagli di spesa si conferma quello degli ultimi tre anni, non siamo affatto sereni. Quanto alle maggiori entrate, le prospettive mi paiono ancora meno confortanti.

Ministeri. Signor Ministro, è come se un padre di famiglia, che a fatica riesce a pagare ogni mese il mutuo, ottenesse un aumento di stipendio dello 0,3 e, invece di utilizzare le maggiori entrate per risparmiare qualcosa o per estinguere più in fretta il debito, decidesse di chiedere un nuovo mutuo, pur sapendo che almeno metà della rata rimarrebbe scoperta. L'altro elemento quasi sottaciuto nelle dichiarazioni ufficiali del Governo è la mancata crescita dell'inflazione, che rimane bassissima pur in presenza di una fase moderatamente espansiva: non è un problemino da nulla, tanto che in Germania ci hanno fatto un'intera campagna elettorale, ma è un tema che meriterebbe più di un approfondimento, perché permanendo questa situazione - un Paese con il nostro quadro debitorio e con un sistema bancario molto fragile non può ignorare i rischi che discendono da una mancata crescita dell'inflazione. Inoltre, colleghi, occorre dire due parole anche sulle prospettive di intervento annunciate per la legge di bilancio. Da ciò che si è compreso, il Governo è intenzionato a presentare una manovra di corto respiro e di scarsi investimenti. Abbiamo appreso in modo frammentario che ci si vuole concentrare sul lavoro dei giovani, sul contratto degli statali, sugli incentivi alle imprese, su famiglia e povertà, il tutto per un intervento di circa 10 miliardi se la serietà con la quale si pensa di affrontare il tema del lavoro è quella con cui in questi mesi sono stati interpretati i dati ISTAT, giocando con i numeri degli occupati, dei disoccupati e degli inoccupati per far credere in un *boom* occupazionale che con ogni evidenza non c'è e non c'è stato, abbiamo poco di cui stare tranquilli. Per non parlare del fatto che si continua a tacere dell'effetto *doping* di una decontribuzione nella quale abbiamo creduto ma che con la sua gestione schizofrenica non ha aiutato né i datori di lavoro a fare una programmazione adeguata della forze da assumere, né tantomeno i ragazzi, che si sono visti proporre un contratto a tempo indeterminato magari in sostituzione di contratti in essere a fini di risparmio dei datori di lavoro - per poi scoprire spesso e volentieri che, finito il contributo statale, di indeterminato rimaneva solo il tempo che sarebbe servito loro per trovare una nuova occupazione. Infine, colleghi, sento parlare di ipotesi di taglio delle *tax expenditures*. Sarebbero ben 468 gli sgravi fiscali da aggredire con tagli orizzontali. Finalmente si parla di fare chiarezza nella selva delle agevolazioni fiscali in cui si disperdono risorse in modo poco proficuo per i cittadini e molto oneroso per lo Stato. Lo diciamo da tempo. Peccato che anche su questo l'approssimazione utilizzata rischia di vanificare quasi tutto. Saremo pure dei gufi - e siamo abituati ormai a essere considerati come tali - ma ci permettiamo di far notare che il taglio dei contributi, non inserito in un contesto di revisione del sistema fiscale, equivale semplicemente a un aumento delle tasse. O questo drastico abbattimento viene viene pensato come misura di copertura all'introduzione di un'aliquota unica, meglio nota come *flat tax*, di cui possiamo evidentemente discutere il livello, oppure siamo di fronte alla solita ricetta proposta dalla sinistra, che recupera soldi pubblici per spendere di più e non per e non per abbassare le tasse. Tagliare le agevolazioni senza abbattere le tasse sarebbe l'ennesimo gioco per camuffare la riproposizione di un'antica formula della sinistra: tassa e spendi, spendi e tassa. queste ragioni, anche a nome dei nostri figli e nipoti, annuncio il voto contrario del Gruppo Federazione della Libertà alla risoluzione presentata dalla maggioranza. Signor Presidente del Senato, un'ultima notazione. Faccio ammenda per non essermene reso conto in Conferenza dei Capigruppo. Ma, dopo che in quest'Aula abbiamo speso giorni interi per discutere di provvedimenti che nella sostanza erano mance e prebende elettorali, ritengo che concedere a un Gruppo undici minuti - comprese le dichiarazioni di voto - sia un fatto lesivo della dignità nostra e dell'istituzione che rappresentiamo.

la riforma degli 80 euro? Peccato che poi si sono viste crescere le tasse indirette, perché, per finanziare gli 80 euro, sono stati fatti tagli ai Comuni e alle Regioni, i tanto decantati enti locali.

le Province sono quasi in dissesto e non riescono a garantire il rifacimento del manto stradale o il riscaldamento nelle scuole.

Se facciamo la compensazione tra numero di lavoratori e numero di ore lavorate, si è addirittura perso lavoro,

Non è questa la verità. La verità è che è aumentata la precarietà. È aumentata la sottooccupazione. Sono diminuite le paghe e stanno calando il reddito *pro capite* e la produttività del sistema.

di persone, vive in famiglie con grave deprivazione materiale. Se guardiamo poi gli anziani, il dato è ancora peggiore. Presidente, forse qualcosa non va. Tutto questo ottimismo e questa euforia non sono

conti, «non va sottovalutata una tendenza che, concentrata sulla ricerca di risultati immediati e quindi su interventi non strutturali, potrebbe generare effetti distorsivi sull'assetto del nostro sistema».

le clausole di salvaguardia, e quindi l'aumento dell'IVA, sono disattivate. Non è vero, perché sono state solo congelate per un anno. Nel 2019 saremo nella stessa identica situazione e l'IVA aumenterà. Ma che certezze hanno gli investitori e le imprese che devono fare una programmazione del loro lavoro, se hanno sempre una spada di Damocle sulla testa, non sanno che cosa succederà e se i loro prodotti saranno concorrenziali o meno? meno? Presidente, serve un'azione incessante e prolungata di riforme strutturali, in grado di ingenerare fiducia, accrescere i tassi di natalità, promuovere gli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali e chiudere il divario di produttività per creare le condizioni affinché gli scenari demografici e economici alla base delle proiezioni siano capovolti.

Signor Presidente, mi auguro che il Governo usi i margini disponibili per fare veramente interventi selettivi e non frammentari, migliorando la qualità della spesa e affrontando le ragioni della bassa crescita del PIL potenziale

Signor Presidente, signor Ministro,

a tutte le leggi di stabilità che portavano occupazione, alle leggi che riformavano il

come ha relazionato in Senato il Ministro dell'economia, hanno portato a quella ripresa economica e dell'occupazione e a quello sviluppo che tutti ci eravamo prefissati; siamo usciti dalle secche di quella che il Ministro ha la più grande crisi dal dopoguerra. Quell'azione ha dato positivi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ovviamente,

Grazie a tutta

idea politico economica che la invitiamo a leggere e che forse potrebbe essere d'aiuto. Noi auspichiamo che il Governo intervenga quanto prima sulla Commissione europea per avere un rapporto sullo stato di attuazione del *fiscal compact*. Com'è noto, tale valutazione preventiva è richiesta dall'articolo 16 del Trattato istitutivo del 2012. Il prossimo anno, in caso di valutazione positiva, all'inserimento definitivo di quelle regole nell'ordinamento comunitario, signor Ministro, un passo denso di conseguenze, destinato a segnare la possibile futura evoluzione dell'economia dell'eurozona in generale e dell'Italia in particolare, di cui lei è il massimo responsabile, responsabile, sia in negativo che in positivo, su questa scelta. Un simile passo non può essere compiuto al buio, senza avere la minima certezza di ciò che ha funzionato e di ciò che, invece, ha contribuito ad aggravare tutti i problemi esistenti. I dati in nostro possesso ci dicono che il *fiscal compact* è stato un fallimento generalizzato. Nessun grande Paese ha rispettato quelle regole, nemmeno la stessa Germania, il cui debito, in rapporto al PIL, doveva diminuire ed invece è aumentato, seppur di poco, anche in Germania. Fa eccezione un certo numero di piccoli sette o otto, la cui popolazione complessiva è inferiore alla metà di quella italiana. Troppo poco per costringere tutti a bere una amara medicina. Naturalmente, nelle nostre valutazioni possiamo sbagliare. Noi non abbiamo, come altri, la verità assoluta. Siamo quindi aperti ad un eventuale contradditorio, che può essere attivato solo dalla Commissione europea, fornendo una serie di evidenze empiriche che consentano un giudizio scevro da pregiudizi. Ma siccome questo lavoro richiederà il tempo necessario, è bene che sia questo Governo e non il prossimo a porre il problema, onde evitare il rischio che l'immediata scadenza della decisione possa fare agio alla preventiva ed indispensabile valutazione di merito. Noi contrapponiamo al «tassa e spendi» i meriti e i bisogni, il che è una rivoluzione copernicana, una evoluzione culturale completamente diversa dall'idea di chi pretende di mantenere lo *status quo* o di ritornare indietro dato che riguarda chi, invece, chiede di andare avanti. Ed è per questo che noi

Articolo 1-MDP voterà a favore dello scostamento dall'obiettivo di medio termine, perché tale scostamento permette di effettuare una manovra meno restrittiva. Lo rende possibile, però, aumentando il disavanzo e quando ci si indebita di più è molto importante scegliere nel modo giusto come impiegare i margini ottenuti. Noi riteniamo che la maggior flessibilità ottenuta negli anni passati sia stata in larga parte sperperata, per questo chiediamo da tempo una inversione di rotta. Siamo molto colpiti dalla lettura rosea che ci propone il Governo nella Nota di aggiornamento al DEF secondo cui saremmo in una fase di crescita economica che si va consolidando, resa possibile dalle politiche fin qui perseguite. Non è così: le politiche fin qui perseguite sono state inefficaci. La relazione della Banca d'Italia del 2017 ci dice chiaramente che l'aumento del PIL italiano dipende per quattro quinti, cioè per l'80 per cento, dalle politiche espansive della Banca centrale europea, il *quantitative easing*, e solo per un quinto

Questa lettura sbagliata degli effetti miracolosi delle politiche sin qui condotte porta il Governo a riconfermare scelte sbagliate del passato, in un'ottica di "continuismo", come la definisce il presidente del Consiglio Gentiloni Noi invece chiediamo discontinuità. Faccio alcuni rapidi esempi. Se confrontiamo la situazione economica attuale con quella di dieci anni fa, cioè con la situazione precrisi, vediamo che il PIL è ancora più basso di allora di 6-7 punti percentuali, che gli investimenti sono sotto del 27 per cento e la produzione industriale del 21,4 per cento. Le difficoltà della nostra economia dipendono quindi, in tutta evidenza, dall'insufficienza del processo di accumulazione; lo *stock* di capitale è insufficiente. La prima ricetta dovrebbe essere aumentare gli investimenti, soprattutto quelli pubblici, che hanno un forte impatto sulla crescita. Invece la Corte dei conti ieri ha certificato che già nei primi otto mesi del 2017 gli investimenti fissi lordi pubblici sono diminuiti del 4,2 per cento rispetto ai primi otto mesi del 2016. Noi chiediamo con forza un'inversione di rotta; per far crescere il Paese e creare occupazione occorre investire di più, in particolare in settori con forte impatto ambientale (dissesto idrogeologico, riqualificazione urbana, efficientamento energetico, eccetera). In secondo luogo, l'occupazione è aumentata ed è prossima a quella di dieci anni fa. Se circa la stessa occupazione di dieci anni fa produce un PIL inferiore del 6-7 per cento rispetto a quello di dieci anni fa, non c'è da essere felici. significa due cose. In primo luogo, molti lavoratori lavorano meno ore; si è infatti registrata, negli ultimi dieci anni, una forte diminuzione delle ore lavorate per addetto

quando va bene a tempo determinato, come ci confermano gli ultimi dati di pochi giorni fa dell'ISTAT, che ci dicono che quelle a tempo determinato rappresentano più dell'80 per cento delle nuove assunzioni. In secondo luogo, l'aumento dell'occupazione avviene soprattutto in settori caratterizzati da una bassa produttività, come il turismo e la ristorazione, e questo deve destare preoccupazione. Aggiungo anche che si tratta di settori con stipendi bassi o molto bassi, che non possono contribuire alla crescita neppure attraverso il sostegno ai consumi, mentre possono purtroppo contribuire alla crescita delle diseguaglianze. L'aumento della disuguaglianza nel nostro Paese non è infatti solo imputabile al forte spostamento del reddito dai salari ai profitti, ma anche al forte aumento della disuguaglianza all'interno del lavoro dipendente, una disuguaglianza dovuta alla forte dispersione dei salari orari e alla crescente differenza nelle settimane e nelle ore lavorate. In questo contesto, ogni misura di flessibilizzazione del mercato del lavoro si traduce in una precarizzazione, come è avvenuto con il *jobs act* e con il decreto Poletti. Quando chiediamo un'inversione di rotta sul lavoro, la chiediamo sulla base di una diversa lettura della realtà economica. Noi chiediamo più tutele sul mercato del lavoro, meno facilità a licenziare, regolamentazione dei finti *stage* e dei tirocini che umiliano i nostri giovani, minore convenienza del lavoro a tempo determinato. Tutte cose che non comportano costi aggiuntivi, ma scelte politiche di discontinuità. Il forte aumento delle disuguaglianze si accompagna all'impoverimento di fasce crescenti della popolazione, in cui si registra una sempre più ampia difficoltà nell'accesso alle cure sanitarie. Noi siamo contrari alla privatizzazione strisciante della sanità e al fatto che si punti sempre di più, per la sanità, sul *welfare* aziendale, pagato da tutti, ma riservato a chi ha lavori continuativi e specialmente a chi lavora nelle grandi imprese. Per questo chiediamo ancora una volta discontinuità, come ricordato dalla senatrice Dirindin, per invertire la caduta della spesa sanitaria sul PIL, a partire dall'abolizione del *superticket*. Scrivere questi obiettivi nelle risoluzioni di maggioranza, come già era avvenuto prima dell'estate per nostra iniziativa nella risoluzione sul DEF, non basta, se non c'è una vera disponibilità del Governo, disponibilità su cui per ora non sono ancora arrivati segnali veri. Per finanziare questa e altre richieste, come il blocco dell'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, chiediamo più determinazione nella lotta all'evasione e abbiamo su questo proposte precise. E invece ci viene riproposto, in continuità con il passato, l'ennesimo condono fiscale (80 in Italia dall'Unità d'Italia in poi: più continuità di così!), che premia gli evasori e beffa i contribuenti onesti. Non ci siamo. Per tali ragioni non voteremo la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento al DEF. Non parteciperemo a questo voto, ma continueremo con forza a batterci per ottenere per il Paese risposte adeguate a questi problemi nella prossima legge di bilancio. È su queste risposte che orienteremo il nostro voto anche a quella legge.

colleghi, colleghe; signor Ministro, ho grande stima per la sua persona e il fatto che lei provenga non da ranghi politici, ma dal dal mondo accademico e dai livelli di competenza che hanno servito la politica, mi ha fatto sperare in un atteggiamento di maggiore orientamento alla verità che deve essere detta al Paese. Temo invece, e lo dico con tutto il rispetto, che il Documento di economia e finanza sia, per così dire, addomesticato alle esigenze politiche e il linguaggio, che ho ascoltato da rappresentanti del Governo e purtroppo anche da lei in questa occasione, non sia orientato a riparare il corto circuito che c'è tra la piazza e il Palazzo. Signor Ministro, sono convinto che il Paese non abbia bisogno di Nembo Kid,

ha ricadute molto pesanti e gravi sui livelli di coesione sociale, debba essere affrontata con un atteggiamento meno orientato ad esaltare i decimali di un miglioramento che non vedo, più che ad impegnarsi a recuperare le ragioni della situazione di grave e perdurante difficoltà e sofferenza economica. che io leggo, nell'esercizio della mia attività politico-parlamentare, vivendo anche nel territorio, nello stato di sofferenza delle nostre aziende, delle nostre imprese e delle famiglie. Lo leggo ancora di più nello stato di grande disagio, disillusione, rabbia, protesta e sdegno dei nostri giovani, quei giovani che non hanno futuro e per i quali non costruiamo una prospettiva

l'estero. Credo che tutto questo emerga nei dati di finanza pubblica, che sono in parte anche esposti con elementi documentali puntuali e precisi nel Documento di economia e finanza. Su di essi, a mio avviso, avremmo dovuto porre maggior attenzione e costruire, a iniziare dal Governo, una riflessione seria

con la copertura in *deficit* della clausola di salvaguardia sull'aumento dell'IVA, che mi sembra soltanto un'alchimia. Così come un'alchimia è celebrare le contraddizioni tra debito e PIL. invece, esplorare l'effetto di ricaduta sulle politiche sociali, su un *welfare* che riduce sempre più le coperture e le garanzie, che produce una condizione di aumento delle diseguaglianze, che riacutizza quelle diseguaglianze che, invece, dovremmo riparare, per restituire un livello vero, pieno e attuato di coesione sociale al patto intergenerazionale che risulta essere gravemente pregiudicato. Tutto ciò al Sud assume colori più foschi e una situazione di sofferenza che si legge nella condizione di maggior e più evidente crisi.

Io voglio bene al Paese, amo il tricolore e vorrei dare un modestissimo contributo e i contribuenti devono partire dal dire la reale condizione di difficoltà in cui si trova il Paese, con una disoccupazione preoccupante, soprattutto al Sud, e una condizione di precariato, che non è solo quello lavorativo: il precariato psicologico è la condizione che mi preoccupa e credo dovrebbe preoccuparci. politiche sociali della sanità mancano risorse adeguate senza il riallineamento tra spesa e PIL e - mi si consenta, signor Ministro e signori del Governo senza il tentativo di dire che forse c'è bisogno di una *governance* diversa nell'ambito delle politiche sociali e soprattutto nella sanità, perché sono convinto che non è cambiando il colore di chi governa il Paese che il problema si risolve. Credo che abbiamo il dovere di dire qualcosa in più su cosa si può fare in termini di *governance* complessiva di una sanità nella quale le dinamiche demografiche e l'evoluzione delle tecnologie portano a uno squilibrio profondo fra la domanda e l'offerta e nella capacità di dare una risposta adeguata

privata dei cittadini. Credo che questi siano gli aspetti dei quali ci dovremmo occupare, insieme alla pressione fiscale che dovremmo contenere più di quanto non si sia riuscito a fare, alla burocrazia bizantina e ossessiva che opprime la libertà d'impresa, al debito pubblico che scende, alle poche parole dette sullo *choc* fiscale di cui avrebbe bisogno questo Paese e alle risorse da destinare al recupero di una politica sociale che ristabilisca uno stato di maggiore coesione tra i cittadini. Credo che tutti questi elementi siano stati affrontati in modo talvolta insufficiente e talvolta inadeguato. Questo mi dispiace. Penso che si debba

sono al riparo da forme di speculazione politica - possano servire a recuperare le ragioni perché nella legge di bilancio si metta un po' di buona

l'aggiornamento che stiamo valutando si fonda su elementi positivi e di assoluto rilievo e - diciamo la verità - fino a qualche mese fa addirittura impensabili. I dati più recenti sul PIL ci permettono infatti di rivedere al rialzo la previsione di crescita del PIL reale, che sarà pari all'1,5 per cento per quest'anno e, probabilmente, anche per il 2018 e il 2019. Sono dati che ci confortano e che testimoniano come le politiche promosse per lo sviluppo economico e il lavoro abbiano cominciato a dare i primi frutti. La nostra è, infatti, una crescita influenzata, oltre che dal buon andamento dell'economia internazionale, anche dall'effetto ascrivibile alla ripresa degli investimenti e al miglioramento del mercato del credito. Inoltre, le prospettive dell'economia beneficiano della rinnovata fiducia degli operatori e del sensibile miglioramento anche del settore del credito, favorito peraltro anche dagli interventi che noi qui abbiamo approvato per riportare il nostro sistema bancario verso una situazione di normalità. L'unico dato macroeconomico che ci preoccupa è quello dell'inflazione e lo diciamo per un Paese fortemente indebitato come l'Italia; inflazione che, però, non cresce anche nei Paesi che stanno meglio di noi, dove i consumi ci sono e dove c'è quasi piena occupazione. E questo è un elemento sul quale, forse, dovremmo tutti riflettere, al di là della maggioranza e dell'opposizione, perché con esso dovremo fare tutti i conti nei prossimi mesi e anni. La strategia del sentiero stretto, cioè tra consolidamento fiscale e sostegno alla crescita, ha consentito sicuramente al Paese di riprendere a crescere e, al tempo stesso, di consolidare i conti pubblici. Il debito pubblico, che pesa sulle prospettive future, ha infatti invertito la tendenza di incremento, che era stato costante tra il 2008 e il 2014. Già nel 2015 l'ISTAT, come è stato detto, aveva registrato la prima flessione. Per il 2017 si stima una riduzione e per il 2018 la discesa al di sotto della soglia del 130 per cento. Indubbiamente, quindi, il lavoro di questi anni ha dato buoni frutti anche sul fronte dei conti pubblici. Dobbiamo, però, evitare il rischio di rimuovere la questione del debito dal dibattito politico contrapponendo l'impegno per la riduzione del *deficit* a quello per lo sviluppo economico e disperdendo così il dividendo

e l'aggiornamento del quadro economico in senso positivo consente di sviluppare politiche in grado di favorire la tendenza positiva dell'economia. Questi dieci anni, avviati dopo la crisi del 2008, che aveva interrotto una stagione di grande ottimismo, hanno inciso in profondità sulla nostra realtà sociale ed economica, sulla vita delle persone e sulla loro percezione del futuro; in particolare, hanno impattato sul vissuto dei più giovani. Per questo sono necessarie politiche che sappiano coniugare investimenti nell'innovazione Grazie a tutta è dedicato questa volta (c'è l'intenzione di farlo) al lavoro 4.0. Dobbiamo infatti incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e promuovere l'occupazione in nuovi settori, prodotti e servizi che ridimensioni la possibile riduzione e la trasformazione del lavoro. Un piano d'investimenti in capitale umano, quindi, è fondamentale per una politica industriale che vuole innovare: investimenti e abbattimento del cuneo fiscale per la produttività, la crescita e il lavoro, ma anche istruzione, rete formativa, alternanza formazione-lavoro, politiche attive d'accompagnamento, servizi al mercato del lavoro sono i principali impegni per il futuro. Esiste poi un altro capitolo sociale altrettanto importante. Negli ultimi due anni in materia di povertà assoluta abbiamo fermato la frana. Questo va detto: il Governo Gentiloni-Silveri ha colmato una lacuna storica del nostro Paese, varando la prima misura anti povertà (il cosiddetto reddito di inclusione). Si tratta di un intervento che debutterà nel 2018, rispetto al quale dobbiamo rafforzare gli interventi e i servizi per sostenere la parte attiva del nuovo strumento. Ben vengano, quindi, le maggiori risorse annunciate dal Governo. Vediamo perciò con favore l'introduzione di strumenti selettivi orientati al sostegno dell'occupazione giovanile, del potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà, degli investimenti privati e pubblici. Per questi ultimi, apprezziamo in modo particolare il fatto che parte delle risorse stanziate anche alle amministrazioni locali, le quali a nostro parere, se virtuose, dovrebbero essere anche destinatarie di misure che consentano lo sblocco e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche. Questi strumenti, a nostro parere, ci consentiranno di sostenere lo sviluppo nelle sue molteplici dimensioni: la qualità del sistema economico, l'integrazione con i mondi della formazione e della ricerca e il *welfare*. Quella che il Governo ci propone, infatti, è una strategia articolata, il cui successo sarà tale nella misura in cui sarà in grado di coinvolgere le istituzioni locali, le imprese, le parti sociali, i cittadini e i corpi intermedi della società;

Per trasformare la favorevole congiuntura in un'espansione di medio-lungo periodo, basata su maggiore innovazione ed equità sociale, necessitiamo infatti di scelte europee di politica economica capaci di favorire gli investimenti pubblici, promuovere le imprese innovative, valorizzare il capitale umano e disegnare efficaci protezioni sociali. Questo significa che, oltre alle politiche monetarie espansive è fondamentale investire sul processo d'integrazione, costruendo, nel contesto della futura evoluzione della *governance* dell'Unione europea, un Ministero europeo delle finanze e una vera unione fiscale europea. Solo con più Europa, infatti, possiamo pensare di affrontare le sfide che un mondo interconnesso e globalizzato ci impone. Nel contesto di un rafforzamento del processo d'integrazione europea, dobbiamo promuovere infatti una riflessione sulle vecchie architetture degli Stati nazionali, valorizzando la funzione delle grandi aree metropolitane, dei territori e delle autonomie locali, che spesso si proiettano nella competizione globale meglio dei sistemi nazionali.

Non ci sarà molto a disposizione, questo è vero, ma quel tanto che ci permetterà sicuramente di camminare a passi più certi lungo questo sentiero stretto che presto, grazie alla politica economica e di bilancio delineata dal Governo, ci auguriamo possa trasformarsi in una strada priva di ostacoli. Il nostro impegno per i prossimi mesi sarà quindi non solo quello di approvare una legge di bilancio che contemperi l'esigenza di non soffocare la ripresa congiunturale con quella di ridurre il debito pubblico, ma anche quello quello di favorire una conclusione positiva e ordinata della legislatura, per consegnare un'eredità forte al prossimo Parlamento e al Paese e non disperdere i risultati raggiunti in questi anni in termini di crescita, riduzione del debito e impegno per l'occupazione.

avevamo registrato la prima vera inversione di tendenza del nostro Paese dopo la crisi economica degli ultimi anni. Nel 2016, il prodotto interno lordo è aumentato, la disoccupazione e le tasse sono diminuite e le riforme strutturali per il Paese erano in corso di approvazione e di attuazione. In altre parole, l'Italia si è rimessa in moto ed è tornata finalmente a crescere. Quello che è stato fatto finora ha rappresentato una fondamentale inversione di tendenza, ma allo stesso tempo non può essere che il primo di una serie di punti positivi per una piena e consolidata ripresa. Siamo soddisfatti delle riforme fin qui attuate, dei provvedimenti di rilancio dell'occupazione e degli investimenti; ma tutto ciò non può che essere uno stimolo affinché Parlamento e Governo continuino sul percorso riformatore. L'operato della maggioranza, sin dal suo inizio, ha perseguito una strategia orientata al rilancio degli investimenti pubblici e privati

assieme all'ambizioso programma pluriennale di riforme strutturali, stanno contribuendo a migliorare la competitività del sistema produttivo. Lungi dal sentirci appagati, signor Ministro, siamo consapevoli che l'anno passato deve costituire la base per un nuovo sviluppo più solido e strutturato, che coinvolga tutti i settori del Paese. La maggioranza e il Governo sono ben consci che gli ostacoli da superare per arrivare a una piena ripresa sono ancora molteplici e radicati da troppo tempo nel nostro sistema Paese. In ogni caso, i dati forniti attraverso la Nota di aggiornamento al DEF 2017 chiariscono che la ripresa economica italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo sia da quelli di occupazione e ore lavorate.

Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8

L'andamento di svariati indicatori suggerisce che il terzo trimestre potrebbe registrare una crescita più elevata rispetto ai precedenti, grazie al dinamismo dell'industria e di alcuni comparti dei servizi, quali i trasporti e il turismo. Le valutazioni delle imprese manifatturiere circa ordinativi e produzione sono ai livelli più elevati dall'inizio della ripresa; il fatturato è già cresciuto fortemente nei primi cinque mesi dell'anno, mentre la produzione di beni strumentali è decollata in giugno e luglio. Anche spingendo lo sguardo oltre l'attuale trimestre, la congiuntura può evolvere ulteriormente in chiave positiva. Il sistema produttivo dovrà essere sostenuto attraverso un rafforzamento della detassazione e dei premi di produttività sulle piccole e medie imprese, da garantire attraverso un medesimo livello di tassazione

per l'orizzonte futuro delineato in questa Nota di aggiornamento, caratterizzata da coraggio e prudenza, determinazione e consapevolezza, innovazione e ponderatezza.

abbiamo espresso anche ieri in conferenza stampa un giudizio molto chiaro sulla Nota di aggiornamento e sulla manovra che il Governo ci presenta.

di dati. La ripresa viene presentata con assoluto entusiasmo, come se fosse interamente frutto delle cosiddette riforme strutturali. Ci chiediamo se è vera gloria. A noi non sembra affatto vera gloria. Signor Ministro, andando a leggere bene tutti i dati, essi sono molto meno entusiasmanti di come vengono presentati, perché si parla - certo - di una maggiore crescita e di una piccola riduzione del debito pubblico,

Per tutti questi motivi, Sinistra italiana voterà convintamente contro la proposta di risoluzione della maggioranza e contro la deroga, non perché siamo per il pareggio di bilancio, ma perché avete sprecato e buttato dalla finestra tutte le risorse che si erano liberate.

a me viene in mente soltanto un aggettivo per definire la recente audizione e le ultime dichiarazioni del ministro Padoan: tragicomico.

insieme all'ex primo ministro Matteo Renzi. Esse non sono scese dal cielo e non le avete ereditate, ma sono il frutto della vostra non politica economica, del fatto che avete trascorso questi ultimi tre anni a fare campagna elettorale a spese

ministro Padoan dovrebbe anche dire che, rispetto al 2008, il monte ore lavorate è sceso di ben un miliardo di ore. Dovrebbe anche dire, il ministro Padoan, che le retribuzioni, al netto dell'inflazione, sono scese del 3,4

di un contratto a tempo indeterminato, grazie al *jobs act*. Anche l'ISTAT ci dice che stanno aumentando i contratti a tempo, per non parlare di quelli di somministrazione di lavoro: precariato su precariato! Il *jobs act* non c'entra assolutamente nulla con questo aumento di occupazione. Inoltre, a parlare sempre di occupazione e di spreco di denari pubblici probabilmente sono diventata noiosa, ma noi siamo gli unici a ricordare che stiamo tornando al punto di partenza, esattamente al 2014. Cosa intendo dire? Avete fatto la decontribuzione, malissimo, che è costata è costata oltre 20 miliardi di euro, a fronte della quale avete stralciato, abolito, abrogato una norma strutturale che aiutava

impeccabile come sempre, la lotta all'evasione fiscale. Voglio parlare di questa lotta all'evasione fiscale, perché sono quattro anni e mezzo che ne sento parlare. Io non mi invento niente, non faccio teorie, esamino i dati

che i risultati del 2016 in termini di lotta all'evasione fiscale riflettono una notevole flessione degli introiti dovuti all'ordinaria attività di accertamento e controllo sostanziale:

fin da quando avete istituito lo *split payment*, che ci sarebbe stata una corsia agevolata per le imprese costrette a pagare l'IVA ai loro fornitori, ma che non la incassano incassano dallo Stato e ne aspettano per mesi e mesi il rimborso. Così lo Stato si può finanziare praticamente *gratis*, invece le nostre imprese, quelle che lavorano con la pubblica amministrazione, sono sempre più strozzate da mancanza di liquidità. Questa è la vostra lotta all'evasione fiscale? Un mero calcolo calcolo contabile a carico delle imprese, quando invece gli accertamenti crollano. Chissà come, non si va a bussare alle porte di qualche amico importante, da cui invece si dovrebbe andare. Si parla, poi, di riduzione del debito.

ora abbiamo sfondato il tetto dei 2.300 miliardi di debito. State qui a chiedere nuova flessibilità, nuovo debito, che sono poi tasse future per gli italiani; ma il problema non è neanche aver fatto nuovo debito: è come lo avete speso, e l'ho detto all'inizio.

No. Noi siamo coerenti con quello che sempre vi abbiamo detto: la vostra politica economica è fallimentare. Il Paese è ancora in ginocchio e la cosa più mortificante è vedere che il *gap* di disoccupazione e crescita tra noi e la media del resto d'Europa, da quando si è insediato Matteo

e lo avete fatto male, punendo gli italiani. Quindi, convintamente voteremo no alla risoluzione e voteremo no all'autorizzazione per lo scostamento, perché per l'ennesima volta si

miliardi di media all'anno, ma già per quest'anno le indiscrezioni ci parlano di poco più di un miliardo, se riuscirete a recuperarlo. Come fanno le aziende a programmare il futuro con promesse che vengono mantenute a singhiozzo?

la registrazione di un'accelerazione della crescita che il Governo annette come conseguenza delle proprie iniziative e, dall'altra parte, un obiettivo di medio termine che nuovamente quest'anno, come negli anni precedenti, viene rinviato. Queste sono le due grandezze da considerare. Cominciamo dalla prima: non nego che

le misure efficaci siano state quelle sul lato dell'offerta: penso alla cancellazione del costo del lavoro sull'IRAP o alla cosiddetta Industria 4.0,

collaborato all'accelerazione della crescita. Qui però sono finite le ragioni di consenso per il Governo e cominciano quelle di dissenso. Nella NADEF non c'è alcun tentativo di riflessione sulle altre questioni, quali è la seguente: la crescita italiana continua a caratterizzarsi per essere inferiore a quella degli altri Paesi europei. Non c'è alcuna riflessione su questo dato. lordo della crescita, se un Paese cresce meno degli altri Paesi europei, si allarga il divario con gli altri Paesi e questo naturalmente si avverte sulle spalle dei cittadini, dei lavoratori e della Nazione nel suo complesso. La seconda questione è che, ovviamente, l'accelerazione della crescita ha beneficiato anche della crescita internazionale. Non vi è dubbio che una parte importante di questa crescita sia dovuta alla componente internazionale.

della volontà e della collaborazione di eventi così numerosi che incidono e producono effetti non voluti all'inizio. Così infatti è stato, a mio avviso: il Governo ha collaborato alla crescita, ma l'accelerazione dipende per buona parte parte da eventi esogeni all'azione di Governo. Questo è importante, anche perché non c'è una riflessione attenta su come rendere strutturale questa crescita. Faccio un solo esempio per ragioni di tempo, ma mi importa sottolinearlo come uomo del Mezzogiorno: il comparto privato più importante del Mezzogiorno è l'agricoltura. Il numero di occupati in agricoltura è enorme rispetto ad altri comparti privati. Non c'è riflessione su questo perché al politico, come credo a tutti noi, dell'accelerazione e della crescita interessano soprattutto le ricadute occupazionali. In agricoltura, per un quadro normativo molto confuso molto confuso e assai penalizzante per certi versi, sia per i lavoratori, sia per i datori di lavoro, si rischia un tracollo. Noi dobbiamo cominciare ad incidere subito su queste materie per fare in modo che quella crescita sia strutturale e quindi incida soprattutto sull'occupazione e sulla condizione dei lavoratori, oltre che su una sana e robusta situazione

Negli anni si è detto che la manovra doveva avere degli elementi temperanti di eventi eccezionali, per alcune circostanze definite in ambito europeo e che queste servivano a consentire di effettuare manovre anticicliche di crescita; invece, questa volta si dice che la crescita accelera, però

interesse che sarà utile considerare nel dibattito, ma qui in Aula la considerazione è politica. A me sembra che l'elemento anticiclico venga violato e questo non ci convince. Signor Presidente, l'ultimo elemento riguarda la questione degli investimenti. Il Ministro stesso riconosce che gli investimenti privati sono ancora al di sotto dei livelli precrisi e che gli investimenti pubblici soffrono. Contraddittoriamente si che bisogna semplificare, ma si invoca il codice degli appalti, che io invece - l'ho detto più volte e lo ripeto - ritengo sia una delle ragioni per cui l'appostazione

quindi nella manovra di bilancio, una riflessione attenta su come ridurre strutturalmente il debito, che è la vera piaga della nostra economia. Per questo, signor Presidente, il voto contrario sulla Nota di aggiornamento e sulla relazione per lo scostamento di medio termine.

ma faccio fatica a capire le ragioni per cui le principali forze di opposizione hanno annunciato il voto contrario alla risoluzione di maggioranza

Vorrei ricordare che l'equilibrio strutturale del bilancio, come è giusto dire in maniera tecnicamente precisa, è previsto non solo dai nostri impegni internazionali, ma dalla nostra Carta costituzionale, quindi è un vincolo costituzionale che abbiamo e la Costituzione stessa, all'articolo 81, afferma che questo non è un vincolo stupido che si applica in maniera ottusa in ogni circostanza, ma deve tener conto delle condizioni del ciclo economico e dei fattori straordinari ed eccezionali. Se ricorrono queste circostanze, il Parlamento può autorizzare il Governo ma, attenzione, lo può autorizzare con una maggioranza più larga di quella necessaria per la fiducia al Governo. Con ciò, in qualche modo, la nostra Costituzione chiama tutte le forze politiche ad assumersi una responsabilità su questo punto. Naturalmente non è obbligatorio per nessuno essere d'accordo con il Governo. Si può benissimo dire che il Governo ha sbagliato a proporre in Europa questo scostamento, perché noi siamo per perseguire in maniera netta e precisa, senza deviazioni, l'obiettivo dell'equilibrio strutturale del bilancio. Io, colleghi, rispetterei in maniera piena chi adottasse questa posizione assumendosi anche la responsabilità di ciò che dice. Faccio più fatica, collega Lezzi (una collega che stimo e con la quale lavoro quotidianamente nella Commissione bilancio),

a sospendere l'applicazione del raggiungimento del pareggio di bilancio e quindi il rispetto dell'indebitamento entro il 3 per cento del PIL», cioè voi proponete un indebitamento sopra il 3 per cento del PIL e dite di no allo scostamento che rinvia di un anno l'obiettivo?

e lo è se ci diciamo le cose in modo corretto, se stiamo ai dati, se non ci attribuiamo cose false, se non diciamo una cosa ad una certa ora e il contrario un'ora dopo, se non diciamo no alla flessibilità che chiede il Governo perché ne vogliamo dieci volte tanto e poi accusiamo il Governo di fare debito facile. Ma la stessa cosa, collega Azzollini, mi consenta, vale per la risoluzione di Forza Italia. Io accetterei la critica da Forza Italia che, come succede, nella dialettica tra destra e sinistra a volte - raramente in Italia perché bisogna ritornare alla Destra storica - incarna la destra del rigore,

impegnare il Governo per un elenco sterminato di spese: maggiore liquidità agli enti locali (e chi può essere contrario), riduzione della pressione fiscale (e chi può essere contrario), misure atte a stimolare la crescita, i consumi e la domanda interna. E ancora: abbassamento dell'età per l'accesso al pensionamento, reinserendo il sistema delle quote e delle pensioni di anzianità

valorizzazione del patrimonio culturale, interventi di prevenzione del rischio geologico. La risoluzione prevede un programma di spese per le quali non basterebbero due bilanci dello Stato.

per denigrarne il lavoro ma l'opposizione è pagata per denigrare il Governo, è pensata per quello. Però distinguiamo tra momento e momento. Certo che ci sono, anche nei documenti dell'opposizione, anche in quello del Movimento 5 Stelle, anche in quello di Forza Italia e in quello della sinistra e di altri Gruppi, spunti interessanti e critici, sui quali un dialogo parlamentare e politico davanti al Paese può essere serio.

se non - ripeto - in presenza di una mozione che dica che essi vogliono e che si impegnano a fare, nella prossima legislatura, politiche restrittive e non più politiche espansive. Se dite questo,

in quel caso di cui parlava un grande dirigente politico, Giancarlo Pajetta, che diceva ai giovani dirigenti politici del suo partito, il Partito comunista italiano (non me ne voglia il presidente Napolitano, magari dico qualche stupidaggine),

so che i miei colleghi non sono cretini, ma sono dirigenti politici, so per certo che non credono alla loro propaganda e allora li invito a votare in maniera seria.

Procediamo alla votazione della proposta di risoluzione Procediamo alla votazione della proposta di risoluzione alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta di risoluzione avrà luogo mediante procedimento elettronico con scrutinio simultaneo.

della percentuale sul PIL destinata alla sanità italiana. Tale percentuale sta scendendo sotto limiti preoccupanti, che vorremmo il Governo si impegnasse a riportare a cifre di livello europeo.

sulla necessità di far passare indirettamente questa legge in determinate condizioni. Ora, quindi, passerebbe il precedente che un partito, un'associazione o un un movimento di qualsiasi tipo attraverso gli insegnanti, in maniera organizzata, utilizzi nella scuola pubblica i suoi aderenti per fare propaganda a quel partito, a quell'idea e a quel movimento. E mi sembra assolutamente inaccettabile. Chiedo pertanto che il Ministero intervenga perché la libertà di insegnamento è sacra. Un singolo insegnante in classe può legittimamente rifarsi alla libertà di insegnamento. Che un'associazione nazionale con 4.000 firme di insegnanti organizzi, invece, in tutte le scuole in cui è presente un coinvolgimento dei bambini su un tema così delicato mi sembra assolutamente fuori posto e chiedo al Governo e al Ministro dell'istruzione di voler rispondere alla nostra interpellanza per evitare precedenti che farebbero diventare la scuola un campo di battaglia.

avermi dato la possibilità di intervenire anche se non mi ero iscritto per tempo. Cogliendo l'occasione della presenza del ministro Minniti, volevo segnalare una questione che riguarda l'importante quartiere Aurora di Torino, dove si sta concentrando, purtroppo, una situazione di tensione legata allo spaccio di droga e alla presenza sempre più massiccia di negozi abusivi. Naturalmente abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale per le sue competenze, ma credo sia necessario un maggiore e più